che mi piace dare a questo intervento è forse apodittico, ma, dopo aver studiato con qualche cura i testi, ripensateci, fermatevi, prima che si perda una grande occasione. Attorno al tema del testamento biologico, più in generale a quella categoria

purtroppo manifestata una sequenza mediatica che ha reso costrittivo un dibattito bisognoso di ben altro agio e di coscienze assai più serene.

di contraddizioni, che certo è vero, come hanno rilevato alcuni autorevoli colleghi, cambia non poco rispetto al primo testo

e non chiude per niente, trasformandoli, i tanti punti negativi che l'opposizione ha segnalato. Si tratta quindi di un suggerimento. Vorrei poi aggiungere che, parlando di argomenti tanto delicati, i quali richiedono il fioretto e non la mazza da baseball, si può incorrere in quello scomodo dilemma che ci sottolineò molto acutamente Rousseau, per cui quasi quasi l'azione morale (perché il nostro dibattito è intriso di questa vocazione, la moralità) consiste in verità nella manipolazione distaccata di norme verso le quali non si nutre alcun impegno personale, se non del tutto astratto. Quindi, tutto questo diventa una forma particolarmente brutale e autoritaria di esternalismo morale, cioè la morale è una sorta di retorica che avvolge testi che non hanno nella coscienza soggettiva più di tanta moralità. Tanto è vero che lo stesso dibattito sulla morte e sulla vita, mi permetterete (da parte

rispetto ad una sorta di tematizzazione rudimentale nella quale qualche volta pare a me di scorgere sembianze perigliose. Dibattito che riguarda la scienza, la tecnologia, perché non sempre le tecniche sono avvolte e governate dalla scienza. Qualche volta - notò un famosissimo informatico, Bill Joy, allora vice presidente di Sun Microsystems - le tecniche più evolute (le nanotecnologie, ad esempio) travolgono le stesse previsioni scientifiche. E un'astratta visione del rapporto tra la scienza e la vita può portarci a questa bizzarria per cui, per un verso, la sofisticazione tecnologica porta con sé armi di distruzione sempre più accurate e, per l'altro, una sorta di appello *post* morale ad una scienza che potrebbe tenere in vita un corpo; ma quale? Il corpo è la sua mente. Un grande biologo, Humberto Maturana, ci ammonisce che la vita è un processo cognitivo. Questo è il grande tema, che nulla ha a che vedere con la religione, la laicità. Altre categorie, evocate con qualche grossolana ubriacatura, anche qui senza offesa per nessuno: non pretendendo di dare lezioni, ma di ergermi qui a coscienza del dubbio prima di affrontare temi così importanti, sì. Cosa c'entra essere laici o religiosi, quando si è di fronte ad una sequenza della storia per cui qualche decennio fa, per uno stesso male, si moriva molti anni prima, ora si muore ad una certa soglia

E il corpo è la mente, se non vogliamo immaginare il corpo una pura manipolazione estetica o, peggio, una tortura. La tortura non è solo quella orrenda che ci viene tramandata da qualche immagine dolorosa, ma è anche una più sofisticata forma di predominio autoritario sui corpi.

dall'opposizione. Ad esempio, cosa ha a che vedere l'articolo 1 del testo con l'articolo 32 della Costituzione, essendo l'articolo 1 una bizzarra riarticolazione di un testo così chiaro? La Costituzione, tra gli altri pregi, ha quello di essere un testo davvero scritto bene, a differenza di questo. Una frase apparentemente innocua "riconosce e tutela la vita umana quale diritto inviolabile e indisponibile" può portare ad ambiguità interpretative del testo. Le leggi sono fatte per essere interpretate è poi l'interprete che decide, non certo l'autore, l'autrice, il collettivo di autori che sta dietro; come per quella definizione - curiosa nella sua reiterazione sua reiterazione - di alimentazione e idratazione, diventati termini simbolici, metaforici, che poco hanno a che vedere con il fatto amaro, drammatico e reale che, a differenza degli altri Paesi, siamo indietro, anche qui, legiferando in maniera un po' bizzarra con un articolato che davvero non va bene. Qualche ripensamento, qualche momento di riflessione sarebbero indispensabili; anche perché c'è da considerare che proprio l'articolo 32 della Costituzione non ci impone alcun dovere di curarci. curarci. La nostra dignità può anche essere questa, ma il testamento biologico, nella sua versione originaria e autentica, significa proprio che ognuno di noi può liberamente scegliere. Lungi da me dare giudizi di ogni tipo su chi ritiene di fare una scelta di fare una scelta piuttosto che un'altra, ma ognuno deve essere, per l'appunto, libero, e guai ad incamminarci in un territorio ambiguo e difficile.

non è etico dare giudizi etici così soggettivi. La salute è un bene primario che ci riguarda da vicino e riguarda la scelta della persona interessata, quando può, con un testamento preventivo biologico serio e rigoroso, con delle banche dati reali (ne abbiamo discusso in Commissione, dove mi capitò di dare qualche contributo spero utile, perché quello della *privacy* su questi dati sensibili poi eventualmente da un consesso che ha, nella soggettività della famiglia, dei conoscenti, delle persone care, del medico, figura rilevantissima ed intellettuale, per così dire mediatore fondamentale in questa vicenda, il punto terminale. Il cardinale Villot, che fu Arcivescovo di Parigi, nonché segretario di Stato di Paolo VI, purtroppo scomparve per un cancro piuttosto cattivo cattivo che lo ridusse in fin di vita con tante sofferenze e disse, proprio prima di spegnersi: «Noi sappiamo dire belle frasi sulla sofferenza, io stesso ne ho parlato con calore. Dite ai preti di parlarne solo per conoscenza diretta. Noi ignoriamo ciò che essa è fino a quando, come è successo a me, non ne piangiamo». Ecco il punto: libertà, diritti, tutela della persona nella sua profonda verità cognitiva di io pensante, ciò che differenzia gli esseri umani dalle altre specie. Ce lo ricorda Stefano Rodotà in tanti scritti fondamentali: il tema che stiamo dibattendo qui non è un tema da poco, e dunque la bioetica, questa nuova disciplina così complessa, non può mai assumere tinte autoritarie o impositive, né può essere un mero riflesso di un'emergenza drammatica, per la quale tutti abbiamo pianto. Guai, dunque, ad ad immaginare queste leggi come normative di eccezione: devono riguardare una nuova soglia della cittadinanza; questa è la sfida che riguarda tutti quanti, qualunque sia la propria religione, laica o credente e quale sia il rapporto con la tecnica, quale sia lo stadio di evoluzione di una civiltà. La persona deve prevalere nella sua complessità e nel suo ruolo fondamentale e quindi, proprio nel quadro delle norme costituzionali sulle libertà della persona e sulla salute, il grande diritto da tutelare è proprio quello che attiene all'autonomia

ma avverso a qualunque scivolamento in tal senso. Ciò che si chiede qui è di tenere conto di una verità che la storia ci ha messo in faccia, proprio per la sua evoluzione scientifica, che tanto distanzia questo periodo da quello in cui si moriva a 20, a 30 a 40 anni, cioè il fatto che noi possiamo, ad un certo punto, avere una nostra autonoma dialettica con la scienza, capire qual è il grado di sopportazione della sua evoluzione tecnica, non esserne succubi e se qualcuno rifiuta, come i testimoni di Geova, di essere trasfuso o se, come è successo anche recentemente, decide che l'amputazione di una propria gamba è un insopportabile guasto della propria dignità, tutto questo va rispettato. Poi si può anche fare l'opposto ed immaginare di poter proseguire la propria vita vegetativa, per così dire naturale, per un tempo lunghissimo, anche attraverso un sondino, ma deve essere una libera scelta. Così è stato anche in altri Paesi e così è in un dibattito che, se spogliato che, se spogliato dalle polemiche di un tempo troppo angusto in cui il confronto invece sta avvenendo ora, se riconsegnato a quella straordinaria opportunità della politica, che è quella di non occuparsi solo della propria quotidianità e sopravvivenza di ceto, bensì del grande interesse collettivo, nel tempo, però, e non solo in uno spaccato limitato e limitativo: cioè la bellezza di poter ergersi a grande teoria della storia. Questo è l'elemento alto della politica: guidare i processi, saperne cogliere la maturazione, non esserne invece subalterni e schiavi. Questo, Presidente, relatore, Governo, colleghe e colleghi, nella speranza che ci si ascolti e che questo Senato, che troppe volte ha subìto la decretazione d'urgenza, persino il voto di fiducia su materie di grande rilievo, sia in questa circostanza, invece, pienamente il Parlamento che legifera, che sa anche interagire, che non prende gli interventi di ognuno di noi come delle pratiche da evadere, come una inesorabile teatralità; sia, invece, frutto di un confronto intellettuale e collettivo, di una voglia di capire che cosa la scelta che stiamo compiendo, quale è il suo grado di mediazione storica. un'altra affermazione forse eccessiva, che però trovo di grande importanza - su questo testo e su questi argomenti, non con una contingenza: dobbiamo invece avere l'ambizione come Assemblea rappresentativa di parlare con la storia, cercando di porvi non un rimedio

mi ha già amabilmente ascoltato in questi giorni durante il lavoro in Commissione. Certo che giunge finalmente in Parlamento una legge importante, che attiene a delle esigenze ben precise, non solo di un personaggio.

Sono in gioco il concetto e la nostra posizione personale sulla vita e sulla morte, su quella fascia intermedia tra due realtà che per noi è sicuramente un aspetto, una dimensione della vita, una fase che comporta debolezza, ma che ha bisogno comunque di aiuto e di carità dando la possibilità a terzi di esercitare questa virtù. Questa mattina e ieri ho sentito parlare di questa fascia intermedia, di persone senza dignità, non persone, non sufficientemente umane. Non so chi possa definire che non sia vita questa fase intermedia. I difensori della libertà, in questo caso magari, assurgono a sostenitori di un comitato che decida chi ha diritto di vivere Ho sentito parlare di stati vegetativi irreversibili. Chi può dire che uno stato vegetativo sia irreversibile? Non sicuramente la scienza. Quindi, la limitazione della libertà può avvenir anche dicendo che queste non sono persone:

mettere in dubbio questo principio, come dicevo prima, significherebbe aprire delle porte pericolose per gli anziani) e la necessità di un'autodeterminazione. A differenza degli altri Stati europei, in Italia si vuole introdurre una legge sul fine vita non basata sulla pietà e sul sostegno di un individuo che sta morendo, ma sul concetto di una libertà che questo individuo avrebbe nel sospendere anche l'idratazione e l'alimentazione. Il relatore sa

costituiti e strutturati dalla società, ma è una libertà dipendente dalla dignità stessa dell'uomo, dalla sua identità, dal suo desiderio, necessità e voglia di vivere. Quindi, libero sì, ma all'interno di una responsabilità che ognuno ha verso la propria famiglia, verso gli affetti e verso regole che, se senz'altro riconoscere la sua specificità di individuo, devono anche riconoscere che questo individuo vive all'interno di una società. Dice l'articolo 32 della Costituzione, che non è mai stato citato, che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.

onestamente per tanti anni in ospedali pubblici, sa quanto i nostri pazienti abbiano il diritto a questa autodeterminazione. In pochi posti come in Italia, a volte, è il paziente ad indicare al medico quale terapia vuole

definire lo stato vegetativo secondo quanto dice il *Clinical Journal of Medicine*: lo stato vegetativo ha delle precise connotazioni e di certo non è un coma. non è un coma. Lo stato vegetativo prevede, come definizione scientifica, un paziente che apre gli occhi, che non ha problemi respiratori e che ha una breve orientazione, sia uditiva che visiva. Quindi, lo stato vegetativo ha una definizione scientifica ben precisa. Per noi questa è vita e, nel dubbio, come ha sostenuto con forza il ministro Sacconi, nessuno di noi può dire che questa non sia vita. l'idea di una precauzionalità si imponga. Il rispetto dell'autodeterminazione può valere solo quando c'è una coscienza e, per gli stati vegetativi, solo per quanto concerne l'accanimento terapeutico, che i Paesi anglosassoni definiscono come terapia stupida e che comunque non va mai praticata in questi casi:

quindi, questi sono trattamenti vitali che sospendiamo, per poi fare un accanimento terapeutico con dei farmaci antidolorifici. Ringrazio, quindi, soprattutto che abbiamo imparato a stimare lavorando insieme in questi giorni, al quale chiediamo ancora un lavoro, che se da una parte tenga sempre fermo il rispetto della vita, dall'altra non si chiuda però su posizioni ideologiche, che non servono a nessuno e soprattutto ai malati e alle loro famiglie.

Vorrei dire che chi mi ha preceduto ieri, e mi riferisco in particolare al senatore D'Ambrosio, ha già messo in luce un aspetto importante, perlomeno per noi giuristi, che ci accostiamo a questa materia in punta di piedi, cercando però di ottenere dalla scienza medica quel conforto che richiederemmo in una sede giudiziaria, facendo una perizia medico‑legale. Non posso credere che la scienza non sia stata in grado di dare un punto di riferimento, quando, rispetto a determinate questioni, l'autorità giudiziaria è stata chiamata correttamente, e correttamente ha deciso, su fatti così rilevanti e si è fidata del punto di vista della scienza. La questione che oggi trattiamo indubbiamente si collega un po' affannosamente al caso Englaro. Mi colpisce moltissimo, peraltro, che mentre il caso Englaro è stato risolto nella sede della giustizia civile, oggi, con il testo sottoposto all'attenzione del Senato, si cerca di spostare moltissimo l'attenzione sotto il profilo penale. Ed è un punto di vista che, secondo me, crea un vizio di fondo, proprio perché finisce con il concentrare l'attenzione su fattispecie

eutanasia, suicidio assistito ed omicidio del consenziente. Devo dire anche che sono rimasta molto colpita dall'intervento del senatore Veronesi, e non soltanto ieri ma anche in precedenza, perché giustamente egli, che per me rappresenta un punto di riferimento - la scienza - ci ha ricordato che ogni legge deve avere lo scopo o di soddisfare le aspettative dei cittadini o di tutelare i loro diritti. Invece, il testo della proposta di legge oggi sottoposto alla nostra attenzione non soddisfa tale aspettativa e soprattutto non tutela il diritto del rifiuto alle cure, tanto che il senatore lo ha definito contro il testamento biologico. Egli ci ha poi ricordato tutto l'*iter* rispetto allo sviluppo del testamento biologico negli ordinamenti del altri Paesi, partendo dall'ordinamento americano, e ci ha anche messo in guardia

un atto importante per un ordinamento giuridico in quanto il denominatore comune è il rispetto e la tutela della volontà di non essere mantenuto in un coma vegetativo permanente. Il cardine e il presupposto di ciò è la consapevolezza che la medicina tecnologica moderna è in grado di spostare il termine della vita al di là della morte naturale, introducendo quindi una vita artificiale a tempo indeterminato, per cui gli organi del corpo umano rimangono vitali anche senza attività cerebrale, in una condizione disumana. il testo che stiamo esaminando non rispetta la volontà espressa dalla persona anzi la obbliga, se in stato di coma, a rimanervi per sempre anche contro la sua volontà, poiché la nutrizione artificiale non può essere rifiutata, in quanto definita sostegno vitale e non trattamento sanitario. rifiutata proprio nella dichiarazione che viene fatta come forma di testamento biologico e questo già pone una forte disparità di trattamento ed un pericolo di incostituzionalità della legge che io, come giurista, sento di dover sottolineare. sottolineare che ho firmato convintamente - lo voglio dire con chiarezza - il disegno di legge presentato dal senatore Marino, perché pensavo che potesse dar vita a una legge saggia ed equilibrata; l'ho firmato quando è stato presentato,

che non lo condivido innanzitutto perché non voglio che il Parlamento emani una legge inapplicabile, inutile, inefficace ed incostituzionale, che dia adito a difficoltà interpretative e sposti sulla magistratura ordinaria o sulla Corte costituzionale

di aver fatto un'invasione di campo, anche se questo è stato poi smentito non soltanto dalla Suprema corte di cassazione, ma anche dalla Corte costituzionale e perfino dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e dall'autorità amministrativa. Se questo è il pericolo che si vuole evitare, il Parlamento sappia che questo testo non lo evita. La proposta, così come formulata, anche dopo l'emendamento del relatore, presenta infatti problemi di incostituzionalità insormontabili alla luce degli articoli 2, 13, 25 e 32 della Costituzione, perché non soltanto si viola il principio dell'autodeterminazione e si annulla sostanzialmente il diritto al consenso informato imponendo dei trattamenti sanitari obbligatori in assenza del pericolo per l'incolumità pubblica, ma la nuova formulazione è in contrasto è in contrasto con l'articolo 25 della Costituzione e i princìpi fondamentali del nostro sistema penale, per la grave indeterminatezza delle fattispecie penali introdotte e l'errata tecnica normativa utilizzata. Si vogliono infatti criminalizzare comportamenti del medico, e anche del fiduciario, allargando in modo generico ed atecnico le fattispecie previste delle norme penali sull'eutanasia, sull'omicidio del consenziente e sull'istigazione e l'aiuto al suicidio - disposizioni , peraltro, impropriamente richiamate in relazione alla materia delle dichiarazioni di fine vita con una previsione non rispettosa delle regole di chi esercita la professione sanitaria, indotto sempre a prolungare la vita del paziente con tecniche artificiali e a tempo indeterminato, anche contro la libera volontà espressa dall'avente diritto. diritto. Norme di difficile interpretazione sotto il profilo dei diritti fondamentali e non tecnicamente adeguate, spesso prevedibilmente viziate sotto il profilo penale, daranno vita perciò ad una legge assolutamente inefficace, che tradisce le aspettative dei cittadini e che, come dicevo prima, farà aumentare il contenzioso giudiziario sia presso la Corte costituzionale che presso il giudice ordinario. Vorrei soffermarmi soltanto su alcuni punti. Ad esempio, dalla lettura coordinata delle norme discende chiaramente che il diritto fondamentale all'autodeterminazione, nonostante il richiamo operato in varie norme del disegno di legge e soprattutto attraverso il rinvio agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione contenuto nell'articolo 1, risulta poi vanificato dalle disposizioni previste da altri articoli. L'articolo 3, comma 6, prevede in via assoluta l'impossibilità di rifiutare l'alimentazione e l'idratazione artificiali e tale disposizione contrasta con il principio costituzionale di ragionevolezza espresso dall'articolo 3; non soltanto perché equipara ai fini della disciplina normativa le diverse tecniche di cui la scienza e la tecnica dispongono e che possono fornire al paziente, ma perché crea quella disparità di trattamento che il senatore Veronesi ha sottolineato. Se infatti una persona in perfetta lucidità di pensiero non desidera più alimentarsi, questa volontà va rispettata, così come sostiene d'altra parte il codice di deontologia medica. Allora, se la volontà di rinunciare all'alimentazione è rispettata quando è espressa in piena lucidità - e ciò si ricava anche dal testo proposto - per quale motivo non deve essere rispettata anche quando è indicata per iscritto e firmata come volontà anticipata espressa nel cosiddetto testamento biologico, senza che questo costituisca una disparità ingiustificata di trattamento che viola il principio dell'articolo 3 della Costituzione? D'altra parte, è anche vero che, così come è configurata, l'esclusione dal possibile contenuto della dichiarazione anticipata di trattamento dell'alimentazione e dell'idratazione artificiali viene a configurare una sorta di ingiustificato trattamento sanitario obbligatorio di dubbia compatibilità con i principi costituzionali. Credo, il caso dinanzi alla Corte costituzionale, la stessa Corte non potrà che riaffermare un'interpretazione costante, e cioè che un trattamento sanitario obbligatorio è sì previsto per legge, ma intanto può essere imposto dalla legge in quanto si

un generico diritto di morire, certamente riconosce su basi costituzionali il diritto al rifiuto delle cure di trattamento, anche di sostegno vitale. La Cassazione ha espresso questo principio consolidato quale principio costituzionale, secondo cui il diritto al rifiuto non incontra un limite nel sacrificio della vita e non esiste alcun dovere di curarsi quale principio di ordine pubblico.

non soltanto della mia parte politica, ma anche della maggioranza, che hanno espresso la volontà di rispettare le scelte della persona e che hanno dichiarato che si asterranno dal votare un provvedimento di questo genere se non ci sarà

che è una scelta di libertà e che corrisponde ai principi costituzionali, la possibilità di compierla, certo non imponendo una scelta di carattere diverso

l'argomento del testamento biologico, come abbiamo potuto vedere dal clamore e dalle divisioni che ha creato nell'opinione pubblica il caso tristemente noto di Eluana, è molto delicato e personale. Ritengo che non sia un ambito dove si possano applicare assiomi validi per tutti e una volta per sempre. Solo individualmente e con la propria coscienza ognuno di noi può prendere la delicata decisione di interrompere le cure in caso di malattie senza prospettive di guarigione, allo stadio terminale, per impedire che le sofferenze o lo stato vegetativo siano inutilmente prolungati attraverso metodi artificiali. Tale decisione non distingue tra terapie, alimentazione o idratazione, ma chiede solo che venga garantito, una volta arrivati alla fine del nostro percorso terreno, il diritto ad avere una morte dignitosa, considerando non dignitose tutte le situazioni in cui le cure mediche non abbiano altro fine che quello di un mero prolungamento della vita vegetativa. Una legge in tal senso, in uno Stato che si dice laico, dovrebbe semplicemente assicurare che le volontà del paziente vengano rispettate, rispettando il suo diritto all'autodeterminazione e a governare la propria vita e la propria morte, come sancito anche dalla nostra Costituzione e come già previsto nel caso del consenso informato. Una legge di questo genere necessita di una discussione la più ampia possibile e della volontà da parte di tutti di arrivare ad un testo in cui non prevalga la visione di una sola parte, sola parte, ad un testo condiviso in grado di rispettare tutti i punti di vista, in cui ogni cittadino italiano, credente o non credente, di destra, di sinistra o di centro, indipendentemente dalla religione dalla cultura o dalle ideologie, possa vedere garantiti i propri diritti. Al contrario, fino ad oggi, da parte di questa maggioranza c'è stato un arroccamento sulle proprie posizioni e la discussione è stata ridotta ad un mero scontro ideologico; alla fine la Commissione ha approvato un testo che di fatto limita fortemente le libertà individuali. Se questo provvedimento sarà approvato così com'è, non cambierà nulla: ci sarà chi continuerà ad andare all'estero per far sì che un proprio diritto venga garantito, o chi sarà costretto ad agire suo malgrado nell'illegalità, come si è rifiutato di fare il papa di Eluana, o chi, nonostante le proprie volontà, sarà costretto a giacere in un letto per anni. Forse servirebbe ricordare a tutti, a tale proposito, la legge n. 194 del 1978 sull'interruzione volontaria di gravidanza, che fu approvata tra mille polemiche. Quella legge, però, ha ridotto drasticamente il numero degli aborti e ha eliminato quasi del tutto il ricorso agli aborti clandestini, garantendo un supporto igienico-sanitario e psicologico alle donne che intendono farvi ricorso. Per molti non sarà stata la migliore legge possibile, ma è una legge che funziona, frutto di una mediazione, e che ha superato gli steccati delle ideologie. Come allora, questo provvedimento non va considerato una conquista sociale, ma la presa d'atto di una situazione che necessita di una regolamentazione, nel rispetto di tutti i punti di vista. Sono cattolica, ma questo non mi impedisce di rispettare le scelte altrui e credere nel principio dell'autodeterminazione. La tecnologia è andata tanto avanti e questo ha avuto implicazioni anche etiche che non potevamo prevedere. Le nuove tecnologie impongono una normativa chiara sul testamento biologico; laddove la tecnologia, la scienza e la medicina non possono più nulla, si lasci fare alla natura e si lasci che quelle povere anime, da tempo in un letto, possano "tornare alla casa del Padre", come fu chiesto ed ottenuto anche da Papa Giovanni Paolo II in punto di morte. Chiedo, pertanto, ai colleghi di mettere da parte l'ideologia e i *diktat* di partito e di votare secondo coscienza, affinché il Parlamento possa approvare un disegno di legge che salvaguardi il diritto di tutti i cittadini a vedere rispettate le proprie volontà.

che non entra nel merito dei problemi. Si è voluto invece rimarcare divisioni, creare confini invalicabili, distinguere artificiosamente tra chi sarebbe per la vita e chi sarebbe per la morte.

non ho mai sentito pronunciare questa parola - e non oggetto della cura. Collocare la persona al centro, renderla soggetto non vuol dire avere un'idea individualistica e radicale della società. Sono una persona di sinistra, la mia storia politica è quella della sinistra riformista, e sono fortemente convinta che il benessere della persona dipenda da un contesto sociale nel quale - oltre ai diritti esigibili - ci sia anche la capacità di esprimere solidarietà.

Nel secolo trascorso, il medico, forte di competenze e di informazioni che erano precluse ai più, ha esercitato sul malato un potere che spesso ha oltrepassato i limiti della libertà individuale, poiché la terapia il più delle volte veniva imposta invece che condivisa. con la scolarizzazione di massa, con l'accesso generalizzato ai *media*, si è assistito ad un progressivo ridimensionamento del potere del medico e su questo mutamento è nata una riflessione, all'inizio degli anni Novanta, precisamente nel 1992,

«è fortemente squilibrato, poiché si stabilisce fra ineguali in termini di competenza tecnica. Orbene, la sensibilità di oggi» - continua il Comitato nazionale di bioetica «vuole riconquistare una dimensione di maggiore equilibrio e anche di equità nei ruoli, esaltando in primo luogo la necessità di fornire un'accurata e analitica informazione al paziente sugli aspetti della malattia, sul suo decorso, sulle finalità del piano di cura proposto, sulle alternative possibili, sulle modalità, sui rischi e sui benefici dei singoli interventi, siano questi diagnostici o terapeutici».

è molto più di una firma apposta per iniziare una terapia, rappresentando la fase finale di un processo informativo che deve essere adeguato alla capacità di comprensione del paziente, il quale può anche rifiutare le cure a difesa della sua integrità psicofisica. di un modello di rapporto tra medico e paziente condiviso, che non significa solo scegliere insieme diagnosi e terapia, ma anche saper condividere, da parte del medico, le gioie e le sofferenze che fanno parte dell'evoluzione di una malattia. Per questo, cari colleghi e colleghe, parallelamente allo sviluppo degli strumenti di autodeterminazione del paziente (quali il consenso informato e le dichiarazioni anticipate), sarebbe necessario far evolvere in modo nuovo la figura del medico. il dibattito in Commissione, ma non mi pare che su questo ci sia la necessaria attenzione. Ai futuri dottori, formati in modo sempre più specialistico, non viene spiegato che il loro compito sarà quello di occuparsi della persona e non solo della malattia:

riproporre qui questioni che abbiamo già accantonato nel dibattito in Commissione sanità? È solo un uso politico per rappresentare in modo fittizio una divisione tra chi dovrebbe essere per la vita e chi dovrebbe essere per la morte? Certamente è un modo per negare il fatto che la scienza medica ha portato uno stravolgimento al concetto di vita e al concetto di morte: quello che prima era un atto naturale, in molti casi è diventato un atto tecnico regolato artificiosamente. Oggi si può vivere per un tempo indeterminato perché le macchine ci tengono in vita, senza che la coscienza, la volontà, le emozioni e i sentimenti, quello che rende il soggetto persona, possa entrare in gioco. Sarà successo a tutti di assistere alla morte di un proprio caro: l'abbandono della vita, se non è inutilmente forzato, è un abbandono sereno ad una morte che ormai non è procrastinabile, per meccanismi tanto complessi quanto dettati da un limite naturale. Chi viene mantenuto in vita artificiosamente non può dire: «Lasciatemi andare», come ha detto Giovanni Paolo

questa legge sarà approvata, metterà in grosse difficoltà coloro che operano nelle terapie intensive e nel settore delle cure palliative, e questo non lo dico io che non sono un medico, ma lo dicono i documenti che ho ricevuto dall'Associazione cure palliative, dall'Associazione dei 2000 volontari che in Italia si occupano del fine vita e da chi opera nelle terapie intensive: nella legge, infatti, non c'è un riferimento al desistere dalla cura quando ormai non c'è più nulla da fare, quando la malattia è inarrestabile e la morte è certa. In quel caso, che cosa è necessario? Desistere dalle cure e intervenire per limitare il dolore e controllarlo il più possibile; inserire inserire il malato in un percorso di cure palliative e, dove possibile, dare un sostegno psicologico e sociale ai familiari.

testo, finanziato a sufficienza, per creare una rete di cure palliative, soprattutto al Sud dove mancano totalmente. Ma sarebbe stato più utile forse tenere insieme tutto il dibattito sul fine vita

in un modo esasperato, quando sono o non sono necessarie alcune forme di sostegno vitale. Ognuno ha portato i suoi argomenti, ma io non penso che in una legge possa essere definito con chiarezza un limite ad una serie di condizioni che sono comunque diverse da persona a persona e che vanno riportate

Sono perfettamente d'accordo, cari colleghi. Ma allora non è un principio di precauzione dire che quando ci sono le condizioni di urgenza e la persona è in pericolo di vita, il medico deve intervenire? principio di precauzione dire che quando la dichiarazione anticipata di trattamento non è più adeguata agli sviluppi delle conoscenze tecniche, scientifiche e mediche, il medico, scrivendolo nella cartella, perché disattende le volontà del paziente, comunque persegue l'indirizzo di di sostenere nella cura il paziente? In tutti gli altri casi pensiamo che la nomina obbligatoria del fiduciario possa consentire di attualizzare la volontà del paziente

di precauzione che abbiamo messo in campo e che abbiamo sostenuto. Abbiamo altresì proposto che fosse il Comitato etico a dirimere eventuali controversie tra fiduciario e medico e che l'obiezione di coscienza fosse altro elemento del rispetto delle diverse condizioni etiche e religiose anche per il medico che deve attuare le dichiarazioni anticipate di volontà. Queste sono forme

parallelo suggerito dal senatore Calabrò tra l'interruzione delle cure a persone in stato vegetativo persistente e i bambini handicappati gravi.

e quindi non può essere fatto un gioco politico sulla pelle di queste persone e sulla pelle di chi crede nei loro diritti. Io personalmente ci credo,

il diritto di essere riconosciute cittadini a tutti gli effetti. Anzi, vi chiedo che questo diritto venga assicurato fino in fondo, sostenendo realmente le famiglie che spesso si fanno carico, in totale solitudine, del gravissimo compito di assistere le persone affette

forzando le loro possibilità economiche, far vivere i loro cari. Avete inserito nei LEA il diritto ad essere nutriti ed idratati,

non c'è stata data, che è stata negativa. Ci auguriamo che alla fine di questo dibattito qualcosa cambi. Il legislatore ha un compito molto importante, quello di consentire l'accesso a un diritto, quello di decidere per chi ha il diritto di poterlo fare soggettivamente, non quello di imporre una scelta. A questo dobbiamo ispirare il nostro lavoro, se non vogliamo che altre sofferenze inutili si consumino sull'altare di un presunto dovere a vivere, anche quando la morte, senza l'artificio della tecnologia, sarebbe un fatto inevitabile proprio per quella che è la nostra essenza umana. *(Applausi

Era diventato una star televisiva, pronto ad essere presente ogni volta che c'era un certo tipo di dibattito e poi, in dieci minuti di intervento, non ha fatto altro che ripetere ciò che aveva già detto

essere stato silurato come Capogruppo del Partito Democratico in Commissione sanità, Morassut per ripagarlo gli ha fatto stampare i manifesti e lo ha fatto parlare ad una manifestazione romana,

perché non sapendosi difendere da solo ha preferito che lo difendesse una collega gentile e brava con la quale mi sono misurato anche in trasmissioni radiofoniche qualche mattina fa. Poteva essere qui a difendere le sue posizioni ed invece è ancora in giro.

avendo vissuto tanto all'estero e avendo preferito svolgere la sua professione fuori dal territorio nazionale tornando poi in Italia con uno pseudobagaglio di uomo infallibile nel mondo della medicina. Finalmente

a migliorare il testo e a compiere tutti i passaggi necessari per migliorare questa legge, come va fatto. È stato un relatore attento che ha seguito l'intero dibattito

come va rispettato un uomo di scienza che ha una sua precisa posizione che noi rispettiamo. Altri, che fanno finta di essere uomini di scienza e invece non

di tutti coloro i quali sono in questo Parlamento, in questo Senato della Repubblica e vogliono migliorare, vogliono riuscire a migliorare il testo del provvedimento compiendo tutti i passi necessari che il relatore Calabrò ha già fatto e che è ulteriormente pronto a fare affinché questa non sia solo una legge voluta dalla maggioranza, ma una legge riconosciuta da tanti e tanti parlamentari che hanno già espresso, prima in Commissione

signor Presidente, si voleva fare di questa legge una passerella artistico-ricreativa, invece di affrontare i temi così come sono stati affrontati da quanti in Commissione, come il relatore Calabrò, vi hanno

che dovete difendere per aver creato quel disastro nella sanità di cui voi siete responsabili. Avete fatto fare solo per pochi mesi al professor al professor Veronesi il Ministro e poi avete preferito non riconfermarlo nell'incarico perché era un uomo libero, che - ricordo - quando

che sono legati al carro della politica e al tentativo di fare di questa legge un'occasione di contrapposizione politica. Sicuramente, con il voto conclusivo del Senato, si dimostrerà che non c'era e non c'è questa volontà, invece, da parte della maggioranza.

intervento, avverto il dovere di rivolgere alcuni ringraziamenti: al relatore, senatore Calabrò, che ha portato avanti il suo impegno con grande e comprovata competenza, al Presidente della 12a Commissione, il senatore Tomassini, che ha saputo condurre i lavori con equilibrio e molto buon senso, al Capogruppo, senatore Gaetano Quagliariello, che ci ha accompagnato in quest'arduo cammino non facendoci mai mancare la sua prestigiosa presenza e i suoi indispensabili consigli, ai commissari tutti, di maggioranza e di minoranza, e sottolineo di minoranza e non di opposizione, che per mesi si sono confrontati su questa legge con passione, a volte mantenendo ferme le proprie posizioni, altre volte cercando e trovando soluzioni condivise, ma sempre nel rispetto delle posizioni altrui, rispetto che un atto così rilevante richiedeva a tutti quanti noi. La proposta di legge che stiamo discutendo e che spero approveremo con ampia maggioranza e con ampia condivisione, rappresenta un passaggio fondamentale e oserei dire storico per la nostra democrazia e per il Parlamento italiano. Come molti di voi in quest'Aula, io ho sempre ritenuto che lo Stato dovesse non entrare nella sfera etica della persona, rinunciando alla tentazione di legiferare in ambiti che competono esclusivamente alla coscienza dell'uomo e della persona. Questo convincimento mi ha sempre guidato in 30 anni di professione medica in terapia intensiva cardiologica, in un ambiente in cui molto spesso, quotidianamente direi, il medico viene a trovarsi di fronte al confine tra la vita e la morte ed è chiamato a prendere decisioni importanti e delicate, quasi sempre da solo, spesso al posto degli altri e del paziente. In tutti questi anni mi ha guidato il senso della scienza, la mia coscienza e, a volte, il buonsenso, tenendo sempre a mente la sacralità, la unicità e il diritto alla vita, ma anche la doverosa dignità nel momento della morte. Il mio convincimento sulla inopportunità di una norma che potesse instaurare o far pensare ad uno Stato etico è stato minato dagli avvenimenti drammatici e dolorosi ai quali inermi abbiamo assistito nell'ultimo anno, e di cui il caso Englaro è stata la testimonianza più eclatante. Il fatto poi che altri, in questo caso la magistratura, si siano sostituiti alla persona decidendo con sentenza, mi ha definitivamente convinto della necessità che dovesse essere il Parlamento, quale espressione della volontà popolare, ad intervenire per colmare un vuoto legiferando in proposito. Questa proposta di legge fissa dei confini ben precisi, partendo da alcuni princìpi inderogabili: certificazione della volontà della persona sui trattamenti medici da accettare o eventualmente rifiutare, nel caso si trovasse nel futuro in una condizione di stato vegetativo permanente o condizione similare; no a pratiche eutanasiche, ma al tempo stesso no a trattamenti che possano mascherare un accanimento terapeutico; conferma della validità dell'alleanza terapeutica tra medico e paziente, soprattutto in un momento del tutto particolare per la persona, che è quello del passaggio dalla vita alla morte; forte ruolo riconosciuto al fiduciario, come garante delle dichiarazioni anticipate di trattamento del fine vita del paziente; conferma che l'idratazione e l'alimentazione, come sostegni vitali, non possano essere oggetto di dichiarazioni anticipate, non essendo nella disponibilità della persona neanche in condizioni di coscienza conservata. Da medico, da laico, mi riconosco perfettamente in questi principi e in questa proposta di legge. Voterò convintamente sì a questo provvedimento legislativo con la speranza, per dirla con il presidente Quagliariello, che nelle strutture sanitarie del nostro Paese da oggi in poi non si debba più morire di fame e di sete.

*(PdL)*. Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, rappresentanti del Governo, con la discussione e l'approvazione del disegno di legge in materia di dichiarazioni di volontà anticipate circa i trattamenti sanitari, il Senato si appresta a dare una risposta chiara su un tema per il quale il legislatore è stato lungamente sollecitato dall'opinione pubblica. Le vicende umane di Piergiorgio Welby nel 2006 e di Eluana Englaro poche settimane fa hanno scosso le coscienze e costretto ad un profondo confronto in seno alla società civile relativamente ai temi del fine vita e più in generale al rapporto tra una scienza e tecnologia medica sempre più evoluta e la salute, cioè la condizione più intima che riguarda ognuno di noi. E' stato un confronto condotto in termini anche accesi ed in qualche caso sterilmente polemici, ma non c'è di che scandalizzarci perché era inevitabile che una questione di tale rilevanza provocasse prese di posizione nette e contrapposte. Posizioni che hanno ciascuna legittimità e dignità culturale e politica ma partendo dalle quali il legislatore deve trovare la forza di fare sintesi, ove possibile, e di fare delle scelte nette, laddove non ci sia la possibilità ulteriore di ridurre i conflitti. In un tema di questa entità e rilevanza, la cosa peggiore sarebbe il varo di una normativa pasticciata ed incongruente in cui, nel tentativo di conciliare l'inconciliabile, si finirebbe per dare spazio alle interpretazioni più svariate, riproducendo una situazione di confusione analoga a quella cui si vuole porre rimedio perché - è opportuno sottolinearlo - l'intento del Parlamento è dettato sostanzialmente dalla necessità

che, ripetutamente, si è pronunciata, anche in sede di giurisdizione volontaria, senza il conforto del diritto positivo. Occorre ribadire dunque con forza che, fino a quando il Parlamento non si sarà pronunciato, non esiste in Italia una norma di legge che consente ad alcuno di condividere, aiutare o favorire il desiderio di una persona a porre fine alla propria esistenza, anche quando la volontà dell'interessato fosse pienamente accertata. È questo un dato di fatto, espresso in modo autorevole anche da esponenti laici (ricordo per tutti il professor Giuliano Vassalli, presidente emerito della Corte costituzionale), che prescinde dalle valutazioni di carattere etico o morale, che inducono tutto un altro ordine di riflessioni sull'argomento. Appartengono a questo secondo filone le considerazioni di quanti ritengono che su un tema così intimamente legato alla vita umana sarebbe inutile e persino dannosa una legislazione dello Stato. Anche questa è una posizione che non si può condividere, perché non tiene in considerazione i problemi posti dall'evoluzione della scienza medica, con il concorso di una tecnologia in grado di penetrare sempre più a fondo in quello che un tempo era ritenuto "il mistero della vita", e che ora, con lo sviluppo della genetica, della bioingegneria, della bioinformatica viene ogni giorno sempre più svelato. La capacità di manipolare la vita umana e le sue stesse basi genetiche è oggi arrivata a tali livelli che l'esigenza di porre norme positive - che sarebbero state ritenute assurde o inutili in un altro contesto - è diventata imprescindibile. Il tema della rincorsa tra avanzamento delle scoperte scientifiche ed elaborazione di un'etica circa il loro utilizzo è già stato ampiamente esplorato riguardo a molte discipline, ma è indubbiamente nel campo della genetica che questa necessità di responsabilizzare i progressi della scienza acquisisce un valore particolare. Per questo non ritengo condivisibile, pur rispettandola, l'opinione di chi lamenta l'invasività di una legge statale sul fine vita, rispetto ad una situazione legata all'esistenza personale di ognuno, perché tale ambito privato è già stato, e viene ogni giorno, violato dalle scelte della scienza e della tecnica. La legge, in questo contesto, non è l'ennesima intrusione del pubblico nel personale della vita, ma ne è la massima tutela. Questa legge ha avuto, come ampiamente prevedibile, un percorso travagliato, che riguarda più di una legislatura quella passata, come ha ricordato il senatore Gramazio, abbiamo già avuto modo di approfondire molto l'argomento). Nel contesto emerso dalla Commissione sanità si denota lo sforzo di tenere conto, fino dove è stato possibile, del ricco e appassionato dibattito svoltosi in questi mesi, accentuato nelle ultime settimane, dopo l'approvazione della mozione conseguente alla vicenda Englaro. Oggi possiamo dire che l'impegno preso dal Senato in quella drammatica situazione non è andato disatteso. Ripugna alla coscienza pensare che la vicenda di questa giovane donna possa essere stato considerato un caso su cui esercitare la polemica politica, ma sicuramente Eluana è stata una lezione per il Parlamento e per il Paese. Nelle settimane in cui si è consumato il suo dramma, l'opinione pubblica ha fatto gradualmente registrare un cambiamento di posizioni. Fin quando la vicenda era percepita come la volontà della famiglia di lasciar morire un paziente senza speranza, la maggioranza degli italiani era parsa favorevole a questo dignitoso decorso, immedesimandosi in vicende che spesso, ahimè, hanno toccato anche le nostre famiglie. Quando però è stato spiegato che la vita di Eluana dipendeva unicamente dal garantire alimentazione e idratazione, cibo e acqua, con un sondino, senza l'ausilio di altre apparecchiature salvavita, il sentimento è cambiato. C'è stato uno spostamento della maggioranza, per come l'abbiamo percepito in molti, verso la necessità di salvaguardare comunque la vita. La reazione emotiva della gente comune è stata *pro* *vita*, questo è un elemento - a mio avviso - indubitabile. Muovendosi all'interno di questo sentimento maggioritario nel Paese, è stata elaborata la proposta che ora perviene all'esame dell'Aula. Una proposta che traccia una linea chiara, discriminante, nel ribadire il rifiuto all'eutanasia, da un lato, e all'immotivato accanimento terapeutico dall'altro, nel distinguere tra quelle che sono terapie e ciò che è unicamente alimentazione e idratazione. L'impegno della Commissione, con un grado di condivisione che è andato oltre le contrapposizioni tra maggioranza ed opposizione, si è particolarmente indirizzato a snellire e favorire l'espressione della volontà anticipata del trattamento sanitario. Sarebbe stato contraddittorio stabilire procedure farraginose o frapporre inutili ostacoli alla libera manifestazione della volontà, considerando che tale *iter* deve poter essere espletato da tutti.

come peraltro si è già parzialmente verificato nell'esame del provvedimento in Commissione. Spiace dover constatare che un tema come quello del testamento biologico sia stato utilizzato dal nuovo leader del principale partito di opposizione, fin dal suo discorso di insediamento, come un elemento per dare una sterzata a sinistra rispetto alla linea seguita dal suo predecessore. È stata questa volontà di riposizionamento, per cercare di porre rimedio all'emorragia di consensi del Partito Democratico, a rendere il confronto di queste settimane più difficili per la maggioranza, con un interlocutore ancora una volta diviso e motivato da esigenze diverse da quelle dell'impegno a dare al Paese una buona legge sul fine vita.

A me pare che la differenza non sia lo scontro tradizionale tra destra e sinistra; mi sembra invece che dialoghino e si contrappongano contrappongano visioni diverse della persona, dell'individuo, del rapporto individuo‑istituzioni ed individuo‑Stato.

ma proprio il tema di fondo del rapporto Stato‑cittadino, in uno Stato che si vuole laico, libero, democratico.

Né mi pare congrua la polemica su chi ha il beneficio di partecipare a dibattiti televisivi, ai quali - lo sottolineo subito, caro collega - avrei voluto partecipare anch'io moltissime volte, se non fosse in vigore sistematico, denunciato persino dall'Autorità garante, a qualunque presenza radicale in qualunque contenitore televisivo. Ci sarei andata volentieri perché questo dibattito non è tra di noi,

E mi appassiona questo dibattito che non trovo, e mi hanno appassionato ed incuriosito una serie di interventi, su cui tornerò. svolgendo sia un dibattito sul concetto della libertà responsabile e della persona, l'essenza della persona. Cosa sarebbe un essere umano privato della libertà

Sono pochi i cardini di uno Stato liberale. Il primo è che il peccato non automaticamente è reato; il secondo è, appunto, che non c'è reato se non c'è vittima.

ed aveva ottenuto anche grandi consensi. Qualcuno ha mutato opinione, molti magari, ma non è un'opinione granitica che sta nella storia. Solo nella legislatura scorsa l'attuale Presidente della Commissione sanità,

Ho sempre pensato, poi, che la Commissione congrua per discutere questo disegno di legge era la Commissione affari costituzionali, perché non è un problema sanitario;

«La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana». Ma lei, signor Presidente, è troppo raffinato per non sapere e non ricordare a cosa si riferiva quella frase

della Costituzione, relativa ai limiti della legge che può determinare trattamenti sanitari obbligatori, ma sempre nei limiti imposti dal rispetto della persona umana. Aldo Moro ebbe a dichiarare, nella seduta della Commissione per la Costituzione del 28 gennaio 1947, dibattendo con un collega forse meno sensibile ad una cultura liberaldemocratica, che quel limite era necessario perché il legislatore non cadesse parole di Moro - nella tentazione dell'onnipotenza, legata - diceva ancora Aldo Moro - a considerazioni di carattere generale e di mala intesa tutela degli interessi collettivi. L'autodeterminazione che può e deve essere temperata da altri diritti, a parte quello del diritto alla vita, a me sembra, invece, che in questa legge venga unilateralmente e totalmente negata. E credo che si sia ricaduti in quella mala intesa tutela degli interessi collettivi di cui parlava Moro. Mi spiego.

disegno di legge afferma, al primo comma, dell'articolo 1, che la Repubblica riconosce il diritto alla vita inviolabile e indisponibile. Ora, se è ovvio che nessuno può disporre della vita altrui, altrettanto ovvio dovrebbe essere il principio che vuole ogni persona libera di disporre di sé, di rifiutare la cura, qualsiasi cura, disponendo intanto della sua vita. Ed è proprio questo diritto che viene, a mio avviso, illegittimamente negato, in particolare quando si vieta al medico la non attivazione o la disattivazione di trattamenti sanitari ordinari sproporzionati alla salvaguardia della sua vita o della sua salute, da cui, in scienza e coscienza, non si possa fondatamente attendere un beneficio per il paziente; scienza e coscienza, infatti, del paziente innanzi tutto non tanto e non solo, del medico o di un legislatore invasivo. In realtà, nei combinati disposti di premessa e poi di normazione, che non si stia introducendo e applicando il diritto alla vita, ma che si stia introducendo un obbligo di vivere, che è un'altra cosa. Dal diritto alla vita stiamo passando all'obbligo di vivere, che contrasta proprio con i diritti fondamentali della persona. È abusivo anche il divieto di rifiutare l'alimentazione e l'idratazione, definite "forme di sostegno vitale fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze", perché mi sembra un'inquietante deriva verso una scienza di Stato,

facendo della sua malattia la più grande battaglia per le cure e per le assistenze anche tecnologicamente avanzate, per rendere sé stesso e gli altri disabili gravi,

C'è per caso qualcuno che pensa di sopprimere i disabili gravi? O pensa lei, relatore Calabrò, di essere il solo a pensare che anche l'esistenza di un disabile grave ha un valore profondo nella nostra esistenza? Pensa di essere il solo?

coloro che hanno inventato una delle frasi più belle, che dovrebbe accompagnarci: dal corpo del malato al cuore della politica. Quindi, vi prego, per onestà intellettuale reciproca, di non tirare in ballo i disabili gravi perché non c'entrano nulla. Così come non c'entra il riferimento a Cameron e alla storia della sua famiglia, né c'entrano i piccoli nati con deficit cerebrali e metabolici. Cosa c'entrano? Stiamo parlando del testamento biologico, cioè del consenso informato di un cittadino adulto del nostro Paese. sottolineo perché è bene che si faccia chiarezza su una serie di vicende che vorrebbero contrapporre un partito della vita a dei fanatici della morte.

questo qualcuno siamo noi. Lo siamo perché abbiamo fato battaglie, anche impopolari, esattamente per

Non ci dividiamo tra destra e sinistra, ma ci dividiamo tra liberali e non, tra laici e non (che è cosa diversa),

In tanti ci siamo domandati se la libertà sia un valore assoluto o non debba piuttosto mirare sempre al bene comune". Ho già evidenziato ieri considero preoccupante il fatto che il bene comune venga prima della libertà individuale, perché lo abbiamo già visto praticare e praticato: non è stata una bella esperienza. Le definizioni dei beni comuni cambiano

è domandati "se l'individuo goda di totale discrezionalità fino al punto di poter decidere della propria vita e del proprio corpo, o se piuttosto non debba arretrare dinanzi al diritto altrui". È certo che deve arretrare dinanzi al diritto altrui, ma che c'entra - ripeto - il disporre di sé con il diritto altrui? Nel disporre di me io non violo alcuno dei suoi diritti; nella sua imposizione, nell'imporre a me e ad altri la sua visione della vita e della scienza, lei calpesta un mio diritto, cioè quello della mia libertà. «se la libertà non degeneri in arbitrio allorché si riduca a cieco egoismo»; e non sia più funzionale al miglioramento del bene personale e sociale». Ripeto: «se la libertà non degeneri in arbitrio allorché si riduca a cieco egoismo»;

che il diritto alla vita non sia l'obbligo di vivere, in particolare se l'ho scritto: non voglio essere attaccata ad un sondino per "x" anni, mesi o settimane. Non c'è motivo al mondo per cui ciò possa essere negato.

Vi rendete conto? Magari nell'emendamento aggiungerete anche il ventilatore, per le ragioni che ho detto prima.

alla libertà di scienza, alla libertà individuale, al rapporto responsabile anche con i propri familiari. E perché mai il medico dovrebbe essere improvvisamente caricato di questa responsabilità?

pensi che l'esistenza di un disabile grave non ha più valore. Guardi, la prego, non è un problema di costi-benefici.

non solo perché non è applicabile, non solo perché è crudele, non solo perché non è compassionevole, ma perché intacca in modo essenziale il rapporto tra cittadini e istituzioni.

onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, fin dall'inizio della legislatura, e ancor più negli ultimi mesi, si è articolato il dibattito sul problema dell'interruzione dei trattamenti sanitari, avendo come obiettivo primario e condiviso la finalità di evitare l'accanimento terapeutico, nella consapevolezza che il limite della vita biologica va coniugato con la sua qualità e con la sua dignità. I punti critici della discussione non mancano. Il confine tra accanimento terapeutico ed eutanasia, la questione dell'alimentazione parenterale, l'obiezione di coscienza, la soglia di condizione di vita considerata accettabile, sono tutte questioni che rendono complessa una regolamentazione normativa e a cui il legislatore deve avvicinarsi con grande umiltà e - direi così - con l'esercizio costruttivo del dubbio critico. Una cosa è certa: in questa materia si ha il dovere di legiferare. Fermo restando che dobbiamo guardare con il massimo di apertura laica al tema dell'indisponibilità della vita, occorre ridefinirne il senso, ma senza ipocrisie. Siamo perciò tutti impegnati alla costruzione di un impianto che, dal punto di vista normativo, possa dare una risposta, non quella unica e perfetta, ma quella, appunto, che più si avvicina ad un possibile equilibrio. Il confronto è aperto anche tra colleghi parlamentari di estrazione culturale e sensibilità diverse, confidando però che si abbandonino - mi deve essere consentito affermarlo toni e riferimenti inutilmente strumentali, tanto più se indirizzati, come abbiamo ascoltato poco fa, a colleghi assenti (peraltro da due ore a questa parte), come il senatore Ignazio Marino, la cui autorevolezza politica e scientifica non può essere messa in discussione, né tanto meno banalizzata. Ricordo che vi sono diverse posizioni anche nel Gruppo di maggioranza alle quali guardiamo, come a tutte le altre, con il massimo rispetto. Ho seguito praticamente l'intero dibattito: fin da ieri pomeriggio nessuno dei miei colleghi del Gruppo del Partito Democratico si è lasciato andare a speculazioni di sorta. È perciò importante, (lo dico al relatore, senatore Calabrò), stimolare e porre attenzione e ascolto alla opinione partecipe dei cittadini e fare in modo che, nelle sedi competenti, il dibattito si sviluppi nel rispetto di tutte le posizioni, nella coscienza chiara e netta della gravità dei problemi e, al tempo stesso, nella volontà condivisa - ciascuno per la propria parte - di costruire una risposta che tenga presenti tutti i valori in gioco. Il legislatore potrà essere molto aiutato da questo confronto ampio nel suo compito, che è quello di trovare una mediazione normativa adeguata. Le famiglie, anche - ma non solo - attraverso lo strumento legislativo, vanno liberate dalla drammatica solitudine in cui versano quando devono affrontare le fasi acute delle malattie incurabili. Scontiamo un deficit strutturale ed anche la migliore legge possibile non può essere di per sé sola il rimedio. C'è il problema della carenza di strutture adeguate per accompagnare dignitosamente nel tempo di vita che è dato di spendere con le cure palliative, ma anche di luoghi convenientemente organizzati per il recupero e per l'intervento a sostegno delle famiglie. A questo tema così delicato ed oggettivamente anche molto impegnativo, l'originaria proposta di legge del senatore Ignazio Marino rispondeva con la previsione di una rete nazionale per le cure palliative, costituita da un'aggregazione funzionale e integrata di servizi distrettuali ed ospedalieri, sanitari, socio-sanitari e sociali, al fine di garantire un'assistenza omogenea su tutto il territorio nazionale, colmando l'estremo divario che si registra - anche in questo settore - tra il Nord e il Sud del Paese. Si è poi stabilito di stralciare questa parte, della quale si occuperà la Camera dei deputati. Non entro nel merito di una decisione già assunta, ma mi sarebbe piaciuto che non fosse smembrata l'idea originaria che mi è parso affrontasse l'argomento nella sua completezza e nelle sue implicazioni di sistema. Do atto al relatore, collega Calabrò, dello sforzo prodotto nel tentativo di pervenire ad una sintesi alta delle varie posizioni e ad un testo condiviso. Tuttavia, devo rilevare che il risultato raggiunto non è pari alle aspettative ed anzi - salvo che non intervengano significative modificazioni in sede di discussione e di votazione degli emendamenti, come mi pare del tutto improbabile - vanifica lo stesso originario intento di legiferare in materia, per le ragioni, che per brevità non ripeto, espresse molto efficacemente da autorevoli colleghi. Alludo, in particolare, agli interventi dei senatori Veronesi, Ignazio Marino, Gerardo D'Ambrosio e Della Monica. Pur nella difficoltà dell'approccio ad un tema così complesso, ritengo utile evitare di soffermarmi su aspetti marginali e cogliere invece la questione più centrale e nevralgica relativa alla nutrizione artificiale e alla idratazione. Lungi da me, naturalmente, la tentazione di addentrarmi in dettagli di natura tecnica, giacché nel mio Gruppo e in questa Camera ci sono specialisti della materia di altissima competenza scientifica, che hanno detto e diranno che che cos'è l'attività integrativa cortico-sottocorticale (ossia l'attività corticale superiore) e che cosa comporta la sua cessazione da accogliere come limite: sostanzialmente questa è la soluzione che l'emendamento Bosone prospetta e che a me pare più che accettabile e condivisibile. E comunque, legando fortemente la modulazione, fino alla sospensione della nutrizione artificiale e dell'idratazione ovvero la sospensione *tout court* del trattamento - alle DAT, giusta l'emendamento della presidente Finocchiaro. Per quel che mi riguarda, ritengo di dover evidenziare brevemente tre aspetti. Innanzitutto, come ho già accennato, la necessità del legislatore di intervenire, ma con la mano leggera, rispettando, oltre che i principi costituzionali e compatibilmente con essi, la volontà anticipata ovvero l'alleanza terapeutica tra medico curante, fiduciario e familiari del paziente (come poi credo che, in larga misura, sostanzialmente si sia sempre fatto). Secondo: le soluzioni prospettate dal mio Gruppo evidenziano un grande, fondamentale rispetto per il bene vita (e per la sua indisponibilità) senza nessun cedimento a derive eutanasiche, ma dicendo no a pratiche di nutrizione/idratazione che, oltre il limite indicato e al di là di questioni astratte, appaiono non più come sostegno vitale, ma sostanzialmente come accanimento terapeutico. Terzo: questa scelta, anche per i credenti, e per i credenti impegnati nell'attività legislativa, deve tener conto dei limiti della scienza e dei rischi di una tecnologia che si sottrae ormai al controllo della scienza stessa - lo segnalava con con forza nel suo ultimo scritto Pietro Scoppola - e quindi può persino risolversi, talvolta in nome della proclamata affermazione dei principi etici, nel loro rovesciamento. La grande tradizione cattolico-democratica è uno straordinario patrimonio, da questo punto di vista, che va reinverato nei mutati contesti di questa fase storica. Vorrei sottolineare che l'esercizio della laicità in politica - nella linea dell'insegnamento di De Gasperi e Moro e di altri grandi maestri che ci hanno lasciato in dolorosa e rapida sequenza negli ultimi anni: lo stesso Scoppola, Ardigò, Elia implica assunzione di responsabilità che va giocata anche con la capacità di mediazione nelle condizioni date in una società pluralistica e complessa. Tanto più quando (come avvertiva ancora Scoppola) queste esigenze e questi valori sono stati variamente interpretati ed espressi in diverse epoche storiche e in diverse civiltà, sicché è impossibile tradurli in un codice definito e permanente di comportamenti. Un banco di prova, al riguardo, sono certamente le questioni che investono la vita dell'uomo, la vita al suo inizio, nella sua fase terminale ma io direi - e qualcuno lo ha ricordato mesi or sono - anche la vita durante, di cui forse si parla meno. I laici credenti impegnati in politica devono essere in grado di esercitare l'autonomia della politica stessa a partire da un'ispirazione alta e vissuta con tutti i rischi, le possibili contraddizioni e incompiutezze che la mediazione storica immancabilmente comporta. E questo ininterrotto esercizio sarà un grande servizio - per quanto ci riguarda riguarda - al Paese e alla sua necessità di inverare i valori nella concretezza storica attraverso il confronto costante che il pluralismo e la complessità culturali comportano. A partire da questa ispirazione ritrovata e da una laicità che sia stile, atteggiamento interiore, direi attitudine "statutaria" del modo di chi è cristiano di stare in politica da cristiano, è possibile riscoprire una grande ricchezza propositiva che incida sulla vita concreta delle persone (la vita durante, come dicevo, innanzitutto) e promuova aggregazione, per quel mondo che condivide quell'ispirazione, ma non solo per esso. Concludo, signor Presidente. L'atteggiamento interiore, con il quale partecipo da parlamentare che fa i conti anche con le proprie convinzioni religiose a questo importante passaggio del nostro compito di legislatori e con cui voterò le proposte del mio Gruppo, è appunto questo: un atteggiamento costruttivo e sereno che spero sia di tutti noi e possa contribuire a soluzioni largamente condivise in cui nessuno voglia affermare per intero il proprio punto di vista, ma tutti concorriamo concorriamo a creare le condizioni di ciò che è il bene possibile. Il bene possibile qui ed ora.

In realtà, penso che sia solo politica, che sia il compito più alto dei Parlamenti, da oggi in poi, perché con la velocità con cui la scienza e la ricerca superano se stesse, di tutta evidenza che questi saranno i grandi temi di fronte ai quali saremo chiamati, impegnati, affinché l'insuperabile, per noi, compito di difesa della dignità di ogni persona sia la guida del nostro agire. Questa legge non è solo finalizzata a redigere norme sul cosiddetto fine vita; è la risposta a "disordini" istituzionali, per cui altri ordini si sono sostituiti e quelli deputati alla tutela della salute. Quando un giudice decide l'obbligatorietà di un farmaco o di una terapia non solo esula dal seminato, ma nuoce gravemente alla salute. Si pensi cosa è stato il caso Di Bella, con un magistrato che ha deciso che quella era una cura adatta. Quante morti anticipate per aver evitato le cure appropriate! Ci stiamo accingendo a pensare, a parlare, e alla fine a decidere, su situazioni che riguardano le singole persone, le loro riflessioni profonde, le loro esperienze personali, le loro concezioni in merito alla ricerca e alla medicina, e sono situazioni che evolvono rispetto alla loro età, al contesto in cui si trovano immerse. Si pensi a quanto si può cambiare una decisione semplicemente, ahimé, in uno stato di grave malattia come la depressione.

È la vita di ciascuna persona che ha valore come criterio per definire qual è il riconoscimento che una società le attribuisce. Nel secolo scorso siamo finalmente arrivati a riconoscere ad ogni individuo uguale dignità e uguali diritti su tutta la faccia della terra e anche chi non ne è consapevole è portatore di questa enorme conquista di civiltà. Su questi assunti l'umanità ha combattuto tutte le disuguaglianze culturali, sociali, sessuali, eccetera; anche il nostro sistema di*welfare* è stato concepito come strumento per rimuovere concretamente, secondo quanto ci chiede la Costituzione, gli ostacoli che ne impediscono la piena attuazione.

Sarebbe un cedimento a scelte ideologiche contraddire questa coerente tradizione, se sostituissimo alla cultura della solidarietà collettiva scelte individuali sul valore della vita. Le norme che ci accingiamo a votare rischiano di andare in questo senso: nel voler fermare in una norma un evento come la fine della vita che non è mai statico, né consolidato una volta per sempre, sia nelle motivazioni individuali che nelle responsabilità deontologiche della medicina che chiede ai medici di ispirare le loro scelte terapeutiche al principio della beneficità

ed è per questo che diffido di chi vorrà interpretare i voti che saranno espressi in Aula come l'OK Corral dei due schieramenti. Non potrei aderire ad un Partito che abbia nel proprio programma scelte bioetiche definitive e non credo che in quest'Aula si aspiri ad avere un partito etico e quindi, ancora meno, uno Stato etico. Il cittadino, e ancor di più il Parlamento, sarebbero espropriati esattamente della libertà di coscienza, fondamento di ogni altra libertà che questa non sia una opportunistica e strumentale scappatoia). Questa legge per molti di noi - ed io certamente tra questi - richiama altre scelte difficili che possono impegnare la coscienza dei parlamentari.

perché in questa sede non solo i cattolici espressero il loro dissenso. Il Paese era altrove poiché sulle grandi questioni etiche il Parlamento può non essere completamente coerente col sentire dell'opinione pubblica perché a questa può accadere che vengano offerte occasioni più di emotività che di profonda riflessione. A noi viene chiesto, invece, di confrontarci, di approfondire, di soppesare e alla fine di deliberare. Questa è la sede in cui si delibera. Personalmente non devo impegnare la mia Chiesa, perché da credente che fa politica impegno solo me stessa, la mia coscienza. Chiedo perciò che dopo l'approvazione di questa legge il Parlamento si senta caricato di un compito aggiuntivo cui non dovrà sottrarsi perché tutti i cittadini che non presenteranno DAT (ed io sarò tra questi) possano contare su un sistema sanitario che garantisce il massimo di assistenza possibile, soprattutto ai meno protetti. Preferisco affidarmi a rapporti di relazione, di cura, tra medico e paziente, a quella relazione speciale e individuale piuttosto che all'automatismo della presa d'atto di una dichiarazione burocratica che rende irrilevante e inficia la responsabilità professionale ed umana. Il Paese ha diritto ad un Servizio sanitario nazionale che da Udine a Lampedusa (soprattutto quando sarà federale) garantisca prestazioni alle cronicità con finanziamenti, strutture, personale di qualità una programmazione di servizi di rianimazione e riabilitazioni, con *hospice* sufficienti in tutto il territorio nazionale coerenti con i dati epidemiologici, altrimenti il resto sono solo parole. È stato detto che 1'eutanasia è superata e ciò perché la terapia del dolore ci ha sollevato dalla insopportabile partecipazione al dolore dei pazienti e dei familiari, ma occorre diffondere di più la medicina palliativa. È un diritto anche questo e il Servizio sanitario nazionale, oltre ad offrirla omogeneamente sull'intero territorio nazionale, deve anche approfondire la ricerca. questo per me è importante la prima parte di questa legge, che conferma il dovere dello Stato a rispettare pienamente la Costituzione, il che, nella sua attuazione pratica, significa un Servizio sanitario nazionale finanziato a sufficienza. Con l'articolo 32 va sempre letta la prima parte dell'articolo 2 della Costituzione, che fa riferimento ad inderogabili doveri di solidarietà sociale. Se ciò non accadrà, dovremo dedurre che Governo e Parlamento hanno solo voluto piantare una bandierina ideologica. Verranno giorni ancora difficili per i parlamentari di tutto il mondo, a causa, come sappiamo, degli sviluppi vertiginosi della ricerca. Dovremo umilmente prepararci con confronti approfonditi e non a rimorchio di eventi mediatici eclatanti, con indicazioni di marcia all'interno di due binari che io vedo necessari: l'indisponibilità della persona e l'intangibilità della specie umana. La domanda di fondo che mi arrovella da quando incominciai ad interessarmi dei problemi umanitari è questa: può un sistema, sia pure democratico, oggi mettere le mani sulle generazioni future? Democrazie forti e ricche decideranno il domani di chi non può né difendersi né tanto meno decidere per sé? Anche il voto di questo provvedimento porta con sé, per quanto mi riguarda, questo tormento. Questa legge ci ricorda che siamo «finiti», che esistono i limiti: nostri e della scienza. È importante saperli riconoscere perché il prometeismo potrebbe condurre all'oppressione da parte del forte sul debole: forte ad ogni titolo, che afferma se stesso con la distruzione della libertà, della dignità, della vita che non considera degna di essere vissuta, perché si arroga lui, il forte, di decidere quale debba essere la qualità della vita che merita di essere vissuta. L'orrore che ne consegue, nel '900 si è manifestato in tutta la sua potenza. Pertanto, partecipo al dibattito con la trepidazione di chi ha la consapevolezza che essere legislatore comporta questa alta responsabilità correlata anche al rischio di sbagliare, sia pure con le migliori intenzioni.

a molti paletti messi dai colleghi, ai punti fermi su temi fondamentali, il mio cuore si è rifugiato in quello che dice Pascal: seguirò quelle ragioni che la ragione, quella che viene spesso invocata come risolutrice di tutto, non può comprendere.

quando il Parlamento italiano ha deciso di normare una questione rilevante nella vita di ciascuno come in questo disegno di legge sul testamento biologico, si sono forse inevitabilmente, e in maniera del tutto erronea, a mio avviso, venuti a creare due schieramenti. In verità, trattandosi di questioni che attengono anche alla coscienza, l'opinione pubblica finisce per dividersi in una contrapposizione falsamente ideologica, poiché temi come la vita e la morte non sono propriamente temi ideologici, ma fanno parte della vita e della morte di tutti i cittadini, qualsiasi sia la loro idea politica. Così ci si contrappone, si discute di quale sia la migliore maniera per disciplinare anche questo momento fatale e si finisce per essere classificati come i cosiddetti cattolici, da una parte, e i laici, dall'altra. Questa spartizione di intendimenti è, a mio avviso, del tutto errata, perché non si deve procedere in quest'ottica: non siamo divisi tra chi vuole salvare la vita e chi la vuole sopprimere, anzi; tutte le problematiche che possono insorgere nella trattazione di argomenti così delicati appartengono soltanto ad una questione di coscienza, in primo luogo, e si collegano alla deontologia del medico e al rapporto di questo con il suo paziente. Sul disegno di legge che siamo a trattare si è detto di tutto e di più, da molti autorevoli oratori in quest'Aula e al di fuori di essa. Io non intendo entrare nel merito di questioni strettamente giuridiche: molti esperti lo hanno fatto e continueranno a farlo. Mi corre l'obbligo, invece, come medico, di approfondire proprio l'aspetto che riguarda la relazione medico-paziente, perché è proprio in questo nodo che si può trovare un'accettabile via d'uscita agli innumerevoli interrogativi che lecitamente tutti - e dico tutti, laici e cattolici - ci poniamo di fronte a scelte così importanti. I progressi della medicina sono sotto gli occhi di tutti ed è innegabile il grande potere che questa scienza ha acquisito nel tempo e probabilmente vieppiù acquisirà. Ma tutti questi devono essere appunto considerati "progressi" finalizzati a migliorare, curare e protrarre la vita umana nel miglior modo possibile. In questo caso la figura del medico diventa piuttosto "ingombrante". Ai medici è stato contestato a volte quasi una certa invadenza di sfere di competenza non proprie fino ad accuse ancora più acerrime, di volersi erigere a giudice che, tuttavia, non può non tenere in conto la volontà del paziente. Uno dei punti fondamentali intorno ai quali ruota il disegno di legge in esame è evitare l'accanimento terapeutico: siamo tutti concordi nel condividere la libera scelta di ciascuno a decidere se la condizione di continuare a vivere solo grazie alle macchine, pur non avendo più una prospettiva di vita, possa essere considerata un accanimento contro la dignità della persona. Parliamo, però, di macchine;

Perseguire la difesa della vita, sempre e comunque, è uno degli obiettivi del codice deontologico cui fa riferimento ciascun medico, come pure non compiere mai atti idonei a provocare deliberatamente la morte del paziente, ma anche rispettare e facilitare il diritto alla libera scelta del malato, tenuto conto che il rapporto medico/paziente è fondato essenzialmente sulla fiducia reciproca e sul reciproco rispetto. E proprio nel rispetto del paziente, il medico deve anche astenersi dall'accanimento diagnostico e terapeutico. E tuttavia, nell'incombenza di uno stato vegetativo permanente, normalmente il medico dovrebbe, dal punto di vista professionale, assumere una rigidità di condotta, ma non di rigore e di princìpi ed a volte di richiami emotivi. Sono almeno cinque le doverose necessità che devo ricordare a me stessa, come medico, e a tutta l'Assemblea: ciascun medico deve essere umile, cosciente, flessibile non sulle regole fondamentali ma rispetto ai mutamenti di rotta che la clinica impone di fronteggiare. La vita, è vero, è fatta di "universali" e di "particolari" espressi dalle situazioni di specie che vanno analizzate sempre considerando la persona che ne è espressione e portatore. Ciò non porta necessariamente al trionfo del dubbio, bensì al suo rispetto, senza l'arroganza e l'alterigia di chi crede di possedere le risposte al di là di tutto. Certamente, il nostro è tempo di lacerazioni e di compromessi. C'è chi ostenta una perentoria certezza dei fatti arrivando a ostentare crudezza e intransigenza; altri, al contrario, ritengono opportuno sostenere che non tutti i compromessi sono censurabili. Parimenti, spesso, tra gli stessi medici, nonostante in chiari princìpi del nostro codice, può sorgere un dubbio che mal concilia la sacralità della vita e la sua intangibilità con la qualità della vita stessa. Da questo dubbio può scaturire una serie di domande incalzanti. Tutte le vite hanno lo stesso valore: l'anziano, il giovane, il bimbo? È lecito sacrificare vite non significative? Quanto è serio il rischio di scivolare sul piano inclinato delle concessioni progressive? Quali sono i mezzi moralmente imperituri? E quando si parla di qualità della vita, dove stabiliamo i limiti delle Colonne d'Ercole, oltre le quali non andare? La vita umana può significare cose diverse: pura presenza di processi vitali senza stati di coscienza; capacità di avere coscienza ed autocoscienza; possesso di tutti gli indicatori di "*human head*" indicati da Fletcher. Come è evidente, le problematiche che ne derivano in senso strettamente medico, sono molteplici. Tutti siamo consci di come l'esercizio della medicina sia mutato in questi anni. Lo si può chiamare progresso ma, al tempo stesso, è una sorta di *deregulation* che mobilita gli esperti di filosofia morale. Ci piaccia o no molti paradigmi sono saltati e, scomodamele, da medici, proviamo ogni giorno ad affrancarci da un "chi me lo fa fare", piuttosto sconfortante e a pensare esclusivamente ad un "per chi si fa", che coglie invece l'esigenza del malato e del prossimo. E questo messaggio morale, insegnatomi molti anni fa è ancora attuale oggi, in tempi in cui le lezioni di etica medica si moltiplicano e molti (se non troppi) sono quelli che le impartiscono, senza chiedersi se i rassegnati ascoltatori riconoscano loro la competenza ed il pulpito per farlo. Non vorrei commettere anch'io questo errore. Molti considerano che il disegno di legge che andremo a discutere presenti limiti morali, deontologici, giuridici. Dopo le due fasi storiche del "prendersi cura" e "curare", da anni se ne è avviata una terza, caratterizzata proprio dalla necessità di allargare e stabilire nuovi confini e limiti. Ma raccogliere nuove indicazioni ed affermare nuovi diritti non deve però trasformare la relazione medico-paziente in un semplice rapporto legale. I nuovi orizzonti che andiamo a tracciare non devono caratterizzare i medici come se fossero una sorta di notai asettici, pronti a ripetere fino alla noia regole paludate paludate e paludose. Per ciascun medico è importante, e questo deve trasparire anche da questo disegno di legge, poter continuare a lottare fino alla morte per salvare ciascuna vita. E qui torna il problema dei problemi: dove è e qual è il limite, a volte impercettibile, che distingue l'accanimento da un impegno curativo? È il paziente ad avere un ruolo centrale nel fissarlo, per l'autodeterminazione che il diritto giustamente gli riconosce? Sarebbe più opportuno, invece, trovare un criterio unitario per indicare una via intermedia tra i doveri del medico ed i diritti del paziente? In relazione a ciò, quale peso devono avere le direttive anticipate di trattamento in un soggetto non più in condizioni di coscienza tali da consentirgli di manifestare validamente un dissenso? Vorrei fare un breve accenno al quadro clinico di un paziente in stato vegetativo persistente, cioè il soggetto incapace preso ad esame in questo disegno di legge. Si tratta di un paziente che è in stato di veglia ma senza coscienza, può sorridere o digrignare i denti, può muovere gli occhi verso oggetti in movimento, ha funzioni cardio-respiratorie conservate, termoregolazione normale. Quanto è irreversibile questa situazione? Talora, un anno dopo l'insorgenza di questo stato, se ne è constatata la risoluzione giudicata a volte miracolosa. Questi presunti miracoli, invece, devono indurci alla prudenza, piuttosto che indurci, senza indugio, a decidere la sospensione di nutrizione e idratazione. Per tutto questo, per i dubbi che ancora abbiamo e le risposte che ancora non abbiamo scientificamente, credo che, alla fine, sia importante ed ineludibile la necessità di salvarsi dalla retorica. Tanto e troppo è stato scritto e detto, ma la retorica non può riguardare i medici, ai quali spetta, invece, di occuparsi, in modo concreto, dei problemi dei malati terminali o dei pazienti in stato vegetativo permanente, come di tutti gli altri pazienti. Ci sono dei punti fermi oltre i quali nessuno di noi, sono certa, intende andare: rispetto della Costituzione; il riconoscimento della vita come diritto inviolabile; il riconoscimento e la garanzia della dignità di ciascun cittadino; il diritto all'informazione; il divieto di ogni forma di eutanasia e la certezza per ogni paziente che, in mancanza di speranza di vita, nessun medico si accanirà sul suo corpo. paziente, va garantito il diritto a scegliere, ad autodeterminare, con il consenso, libero e consapevole, ogni tipo di trattamento sanitario cui intende o non intende sottoporsi. Il progresso ci ha consentito di migliorare le condizioni di vita e, in termini di civiltà, non possiamo oggi arretrare condannando a morire di fame e di sete una persona solo perché per mangiare ha bisogno di un intervento esterno. Sarebbe come condannare un disabile, un anziano e tutti coloro che comunque non sono autosufficienti. La scienza ha lavorato tanto, con il sacrificio ed il contributo di molti, per arrivare ai risultati odierni in tema di salvaguardia e miglioramento delle cure, e tutti abbiamo salutato questi progressi come segno di civiltà e di modernità. Non cancelliamo le conquiste fin qui ottenute, non cancelliamo i successi ottenuti, ma adoperiamoci per continuare ad offrire a coloro ai quali, sfortunatamente, il destino ha riservato una sorte avversa, la possibilità di continuare a vivere, se lo avranno stabilito, finché vita sarà,

Quindi, è bene che ci impegniamo a modificarlo ed a ragionarci. Il nostro Paese aveva bisogno di una legge sul fine vita e noi ci proponevamo di pervenire ad un provvedimento che potenziasse tutto l'*iter* del consenso informato,

una legge che fosse uno strumento utile, agibile e fruibile da tutti i cittadini: quei cittadini che decidessero, non per obbligo ma per scelta, di governare il processo della propria morte (della propria, non di quella altrui), quando la ragione svanisce e l'io cosciente soccombe ad una vita solo vegetativa, che tale può protrarsi per un tempo molto lungo, quando il confine fra le cure intense e l'accanimento terapeutico per malattie irreversibili ad esito infausto è difficile da rintracciare. Si tratta quindi di governare il processo della propria morte, perché questa è la legge sul sul testamento biologico, in alleanza terapeutica con i medici, con l'aiuto delle persone care, per allontanare il dolore ed allontanare, da coscienti, la visione di un sé in balia della prigione tecnologica e medica inutile ed impietosa. Il

pesantemente su tali diritti di terza o quarta generazione, dicendo: "Se volevate questo, dovevate riscrivere la Costituzione". Non è affatto vero: c'è una dottrina costituzionale molto diffusa che afferma che i diritti di terza e quarta generazione siano tutti compresi e rintracciabili nell'articolo 2 della Costituzione italiana, che è finestra, via e veicolo importante per individuare e normare anche tali diritti. Ha ragione dunque la presidente Bonino: questa è una discussione eminentemente costituzionale. Quando parliamo di diritti di quarta generazione, non accenniamo a nessun titanismo o prometeismo, ma solo all'esercizio umile, doloroso ed estremo della propria libertà quando la fine si avvicina, dell'uso del proprio corpo, come lo si vuole, come lo si percepisce, insomma del proprio ultimo esercizio di autodeterminazione. Arrivati a questo punto, è legittimo è legittimo chiedersi: era proprio necessaria una legge? Eravamo in grado di affrontare il livello della legge? Lo eravate voi come maggioranza? O aveva ragione il professor Veronesi ad indicarci ieri l'esempio tedesco piuttosto che le altre legislazioni di tutto il resto d'Europa e dei Paesi anglosassoni? Aveva forse

il quesito se non fosse legittima anche un'altra strategia: una volta intrapresa la via della legge, bisognava sapere che in essa è insita la nozione di compromesso attivo, di buon compromesso, così come fu per l'aborto, per giungere ad una soluzione legislativa che trovi la condivisione sostanziale del Paese e del popolo, non soltanto delle borghesie colte e dei ceti intellettuali; una confluenza reale tra mezzi e fini, una buona legge che servisse. Il disegno di legge che il relatore Calabrò ci ha consegnato, come hanno sottolineato moltissimi colleghi, crea più problemi di quanti ne risolva, ed esorto a non sottovalutare la prima valutazione dei medici italiani: ha evidenti profili di incostituzionalità; dice troppo e troppo poco; in genere, dice male.

nel tunnel di una confusione proibizionistica il ruolo del medico e i suoi compiti e gettano l'autodeterminazione terapeutica del paziente in balia di mille discrezionalità, di conflitti, di aleatorietà: troppi conflitti in certe soluzioni. Dunque, perché questo è avvenuto? Secondo me, ciò è avvenuto perché, dall'inizio alla fine, il Popolo della Libertà, in tutte le sue sfumature, talvolta ha cercato di fare uno scontro ideale di princìpi esplicito, talvolta insidioso, sotterraneo. Ma questo è avvenuto perché, fra tutte le casistiche di principi di cui abbiamo parlato, il PdL, la maggioranza, non ha mai accettato la prospettiva che, anche di fronte a cure non sproporzionate (l'essenza dell'articolo 32 della Costituzione), il paziente potesse rifiutarle. Questo concetto di autodeterminazione consapevole non è mai stato accettato, accolto, introiettato culturalmente, vissuto. Questo era il *terminus a quo* da cui partire per costruire la soluzione di compromesso, invece è stato esplicitamente e ideologicamente combattuto, senza fine. senza fine. Noi dovevamo contemperare due principi, l'autodeterminazione del paziente e i valori della vita, la cura sempre, quando la si vuole, la sollecitudine estrema, specialmente per i soggetti più deboli, sempre se la si vuole. Questi due principi, però, dovevano essere messi in armonia fra di loro, non una frontale contraddizione dall'inizio alla fine. Lo sottolineo: dall'inizio alla fine. Ecco perché, allora, avete potuto montare questa storia dei malatissimi, dei malati gravi, degli handicappati, degli abbandonati. Ma quando mai? mai? Il problema che non è stato accolto, neppure sfiorato, neppure capito, è che la Costituzione italiana difende ogni individuo come fine a sé, protegge la persona costituzionalmente, la persona che non è strumentalizzabile a fini collettivistici, né sacrificabile in nome degli interessi generali. E, quindi, la rinuncia consapevole ad una terapia non può essere limitata per ragioni sovraindividuali, perché è un diritto costituzionalmente garantito alla cui concreta attuazione il medico è legittimamente chiamato a contribuire. E se non è questo, allora l'alleanza medico-paziente diventa una gabbia. E se non è questo, allora l'alleanza medico-paziente diventa il potere indiscriminato del medico. E se non è questo, allora,

non da tutelare e da rispettare, perché allora avere espresso delle volontà sul sé, anche quando in stato di essere moribondo e pure nella condizione di moribondo, va riconosciuto come persona con piene capacità, perché quando era pienamente persona aveva deliberato su di sé. Questo è stato il problema. In qualche caso noi abbiamo combattuto in Parlamento un grande confronto concreto sulla legislazione, sui valori, sull'autonomia della politica quando suggeritori esterni di varie funzioni legittimamente esprimevano le loro opinioni, ma meno legittimamente ci inviavano gli emendamenti.

da affrontare con umiltà, senza le fiaccole della verità, ma con il lume tenue ma sicuro della propria libertà e della propria autodeterminazione. In conclusione, voglio riservare un pensiero rispettoso al signor Englaro che con la sua straordinaria forza ha potuto, durando (perché la forza morale è grande quando dura, quando non è espressione di un momento), dare una consapevolezza nuova a questo Paese che affronterà, io credo con maturità, i problemi che ha di fronte

signor rappresentante del Governo, nel dibattito sul testamento biologico che si sta svolgendo in quest'Aula semideserta bisognerebbe - come anche affermato dal Presidente di questa Assemblea - mettere da parte le diverse visioni politiche per risolvere un problema che lascia ciascuna coscienza divisa e incerta, qualunque sia la decisione che ritenga giusta. L'immagine di Eluana, qualunque siano le convinzioni personali di ciascuno di noi, ci angoscia rimanendo davanti a nostri occhi. La domanda che bisognerebbe porsi laicamente, al di là delle convinzioni politiche, ideologiche, religiose, è la seguente: "può una persona adulta, in grado di intendere e di volere, nel pieno delle sue facoltà mentali affermare che in caso di incidente grave, piuttosto che rimanere per tutta la vita immobile su di un letto, preferisce morire, invitando chi gli sta intorno ed i suoi cari ad eseguire questa sua volontà? Non è un caso di eutanasia. Semplicemente non bisogna infierire sul malato, e lasciare che la natura segua il suo corso". Come è avvenuto per Horst Tappert, l'attore tedesco che interpretava il popolare ispettore Derrick, deceduto lo scorso 13 settembre all'età di 85 anni in una clinica di Monaco di Baviera come ha detto la moglie Ursula, raccontando che il marito aveva firmato il testamento biologico - i medici, su indicazione della moglie, hanno rispettato l'atto scritto, eliminando la flebloclisi e staccando la spina per la respirazione artificiale quando le condizioni dell'attore sono diventate disperate. «Voleva vivere con dignità. L'ho lasciato morire. Quando ho visto che le sue condizioni peggioravano di giorno in giorno, che non riusciva a parlare e che non aveva più percezione di nulla, e che quando prendevo la sua mano non la sentiva, ho consegnato ai medici curanti il testamento biologico, che avevamo firmato insieme alcuni anni fa», racconta la moglie. Tappert era malato di diabete in forma grave e il suo stato era andato peggiorando rapidamente negli ultimi anni, fino a costringerlo su una sedia a rotelle. «I medici hanno tentato di salvarlo fino all'ultimo. Mio marito amava la vita, ma voleva vivere in piena coscienza e dignità. Abbiamo dovuto constatare che ormai tutto era inutile e ho deciso di rispettare le sue volontà. Temo che adesso le mie rivelazioni faranno scandalo e scateneranno un'ondata di proteste, ma io non ho dubbi. Nessuno può essere costretto a sopravvivere in condizioni inumane. Ci sono pazienti che vengono tenuti in vita artificialmente. Grazie ai macchinari il cuore batte e i polmoni respirano, per anni e anni. È solo apparenza. Non bisogna rimanere vittime di una pratica così crudele». Nel dialogo sulla vita con il cardinal Martini, il professor Ignazio Manno citava il catechismo: "L'interruzione di procedure mediche onerose, pericolose, straordinarie o sproporzionate rispetto ai risultati attesi può essere legittima. In tal caso si ha la rinuncia all'accanimento terapeutico". Giovanni Reale, un grande nel mondo della filosofia cristiana, ricorda: "Attenzione, così non si vuole procurare la morte ma si accetta solo di non poterla impedire". E quando gli si chiede ancora perché, se la vita è sacra, si può pensare di staccare la spina, il filosofo credente mette in guardia dalle insidie di una tecnologia troppo potente che fa oggi dell'uomo una cavia impotente. «Il rischio è trasformare la sacralità della tecnica nella sacralità della vita. E fare fino a dove si può fare all'infinito». Prima di dire di qualcuno che è felice, bisogna aspettarne l'ultimo giorno. Così, più o meno, scrivevano Ovidio, l'autore delle "Metamorfosi", e tanti sapienti antichi. Premeva loro di avvertire gli umani cui sembrasse arridere la fortuna: non se ne sentissero al sicuro, e gli altri non li invidiassero, fino all'ora della morte, e anzi alle esequie avvenute. Montaigne cita Plutarco: a uno che invidiava il re di Persia, arrivato così giovane su un trono così alto, lo spartano Agesilao rispose «già, ma nemmeno Priamo era stato infelice a suo tempo». In una recente intervista Giovanni Reale, vedeva nel caso di Eluana Englaro un abuso da parte di una civiltà tecnologica totalizzante, così gonfia di sé e dei suoi successi da volersi sostituire alla natura. Si è perduta la saggezza della giusta misura. La Chiesa, e il Governo insieme a lei, sono vittime di questo paradigma culturale dominante. Racconta di sua madre: «Era all'ospedale con il cancro, i medici volevano riempirla di tubi. "Potremmo prolungarle la vita di qualche mese", dicevano. Io ero frastornato. È stata lei a decidere: "lasciatemi morire a casa, nel mio letto". Quando Socrate deve bere la cicuta, qualcuno gli suggerisce: "C'è ancora qualche ora, attendi finché il sole non sia tramontato". Ma non ha senso aggrapparsi alla vita quando ormai non ce n'è più. Se mi trovassi nella condizione di non aver più speranze di guarigione», aggiunge Reale, «non avrei dubbi su cosa scegliere». Reale, da credente, oltre a rivendicare la libertà di coscienza dei cattolici, afferma che questa è un preciso dovere morale, senza lasciare alcuno spiraglio all'eutanasia. Non dice "fammi morire", ma "lasciami morire come ha stabilito la natura": né io, né tu, ma la natura. Prendiamo il caso di Piergiorgio Welby, che aveva seguito da vicino. Welby sostanzialmente non disse di staccare la spina, ma disse: "Lasciate che la natura faccia il suo corso, non fatemi restare vittima di una tecnologia che costruisce qualcosa di sostitutivo e di artificiale rispetto alla natura". È un'affermazione identica a quella che si dice abbia fatto Giovanni Paolo II: "Lasciatemi tornare alla casa del Padre". Il secondo aveva fede, il primo no. Per Welby era andare nella notte assoluta, per il Papa nella vita, ma dal punto di vista umano è la stessa condivisibile richiesta. La questione fondamentale che si pone, alla quale si deve dare una risposta, non è quindi l'eutanasia, ma il riconoscimento del diritto di una persona di far valere la propria volontà, a condizione che questa sia stata espressa in maniera chiara ed inconfutabile con l'affermazione di non voler continuare a vivere in stato vegetativo. Si deve stabilire se il diritto che viene riconosciuto ad una persona cosciente di rifiutare le cure mediche o l'alimentazione scompaia quando la stessa sia in stato di incoscienza. La volontà dell'individuo, pur con le opportune garanzie, deve prevalere su tutto il resto. È la visione laica propria di uno Stato moderno che basa i suoi princìpi fondamentali sulla democrazia liberale e sul rispetto. Amedeo Bianco, presidente dell'ordine dei medici, rileva che il 55 per cento dei medici considera pessimo questo disegno di legge sul fine vita, aggiungendo che tutte le comunità scientifiche sono concordi nel ritenere nutrizione ed idratazione obbligatori come trattamenti sanitari, non come forme vitali di sostegno. "Di lì, avvolto nel suo mantello dorato, se ne andò Imeneo per l'etere infinito, dirigendosi verso la terra dei Ciconi, dove la voce di Orfeo lo invocava invano. Invano, sì, perché il dio venne, ma senza le parole di rito, senza letizia in volto, senza presagi propizi. Persino la fiaccola che impugnava sprigionò soltanto fumo, provocando lacrime e, per quanto agitata, non levò mai fiamme.

Proprio per evitare altri casi Welby ed Englaro, simboli delle battaglie per il diritto degli individui all'autodeterminazione, bisogna votare una legge rispettosa degli uomini e delle donne che la cultura dell'intolleranza e della faziosità vorrebbe impedire. che sia travalicato il diritto naturale degli uomini ad una morte giusta e naturale, che la tecnica abbia il sopravvento sulla volontà espressa; si deve ritrovare quella dimensione umana per impedire di costruire uomini bionici, tenuti in vita artificiosamente allo stato larvale privi di coscienza ed identità, ma ben funzionali al paradigma dottrine ecumeniche deviate racchiuse nello spiritualismo. Proprio in questo momento di profonda crisi economica, sociale e di valori, bisognerebbe praticare l'unità. Chi afferma di amare e rispettare la vita non può imporre agli altri la propria volontà, non può sconfinare nel libero arbitrio, costringendo uomini e donne a vivere in condizioni disumane.

Desidero innanzitutto ringraziare Beppino Englaro, che ha fatto una grande battaglia. Se oggi siamo qui, lo dobbiamo in larga parte alla sua azione.

ha costretto tutta la comunità nazionale, l'opinione pubblica, le famiglie ad interrogarsi sul fine vita. Beppino Englaro ha rifiutato fin dall'inizio la classica ipocrisia italiana

Speravo che, dopo il clamore provocato dalla morte di Eluana e lo scontro che si avviò nel Paese tra presunto partito della vita e presunto partito della morte,

quello scontro ideologico purtroppo non si è attenuato. Era bene riflettere e non farsi prendere la mano, era bene prendere del tempo aggiuntivo, invece si è voluto accelerare l'approvazione di questo provvedimento,

che raggiungesse una sintesi elevata tra le diverse sensibilità di questo nostro Paese, tra chi crede nella sacralità della vita e chi ha una visione laica di essa.

che oggi incidono solo sul nostro Paese: da un lato, la posizione cosiddetta teocon, di emanazione americana, che arriva sempre in ritardo in Italia, e dall'altro lato l'influenza delle gerarchie cattoliche vaticane,

della vita, dei vincoli, dei limiti che a mio giudizio non possono essere posti. Avremmo dovuto costruire un provvedimento che fosse la sintesi massima

Quando c'era la vecchia Democrazia cristiana, ci sono stati scontri formidabili sulle vicende del divorzio e dell'aborto. La Democrazia Cristiana, che era un partito cattolico, chiaramente si oppose in Parlamento, ma consentì che quei provvedimenti

invece, con questo provvedimento, costruiamo un modello veramente pericoloso, a cominciare dall'interpretazione che viene data sul tema dell'inviolabilità e dell'indisponibilità della vita:

ha creato delle psicosi nell'opinione pubblica nazionale, perché togliere l'acqua, il pane o la carne ad una persona sembra una cosa che non è di questo mondo, invece in quel caso

Dall'altro lato, si dà un potere ai medici di smentire quando vogliono, attraverso obiezioni di coscienza e valutazioni mediche, ciò che un paziente dichiara come sua volontà sul fine vita,

sarà ancora molto aperta, nel senso che a mio avviso, se verrà approvato un provvedimento in contrasto con la storia laica e liberale di questo Paese,

la stessa fine che fece Fanfani quando volle promuovere il *referendum* sul divorzio, spinto dalle gerarchie cattoliche vaticane. Raccolse le firme e iniziò quella battaglia. Poi, quando andò in giro per i paesi dell'Italia, si accorse che tutta la rete ecclesiale e anche molti parroci erano a favore del divorzio, così come sono stati a favore dell'aborto. Ci furono poi quei risultati formidabili, che segnarono l'inizio della crisi della Democrazia Cristiana. Non voglio che questo succeda al PdL: c'è ancora tempo per fermarsi e ragionare; c'è ancora tempo per costruire un provvedimento condiviso e liberale su cui si possano riconoscere tutti. Se si andrà avanti su questa strada, che considero profondamente sbagliata, sono convinto che ci troveremo tra molto tempo in una situazione analoga a quella in cui si trovò Fanfani.

Vi è una contraddizione nel modo di procedere dei lavori di questa Assemblea parlamentare. Più e più volte si è ripetuto che sul cosiddetto testamento biologico non erano vincolanti le posizioni di partito. Invece, la libertà di coscienza, anima e sostanza di un confronto senza pregiudiziali, appare un dato estrinseco e residuale. C'è piuttosto una linea da far valere, anzitutto sul confine tra maggioranza e opposizione. A tal punto che il Presidente del Consiglio indica alla sua maggioranza la strada da seguire, a dispetto di ogni precauzione circa l'opportunità, se non altro, di mantenere il Governo su un piano di corretta e prudente neutralità. Può essere l'Esecutivo a stabilire cosa fare su una materia come questa, che implica o dovrebbe implicare l'assoluto rispetto delle posizioni e delle scelte dei singoli parlamentari? Certo, così non dovrebbe essere e così per contro si vuole che sia. Si pretende di fissare una demarcazione anche in un ambito in cui vige il primato incontrovertibile della responsabilità personale. Avevamo sperato che il bipolarismo non dovesse implicare la divisione radicale sulle questioni dell'etica e della biopolitica. Indubbiamente tra centrosinistra e centrodestra vi saranno, oggi o domani, anche in questo campo differenze significative; ma nessuno può e deve escludere che in alcuni casi subentri una ragione condivisa o una convergenza su punti qualificanti. Non è detto che il Paese si rispecchi solo nella fredda e lucente fotografia delle rispettive angolazioni dottrinarie, più o meno filtrate attraverso una riserva di pubblica tolleranza. In un passaggio emotivamente carico di tensione, all'indomani della morte di Eluana Englaro, alcuni di noi hanno ritenuto giusto approvare il dispositivo della mozione che la maggioranza aveva presentato come atto d'indirizzo in vista, appunto, della redazione del testo di legge ora all'esame dell'Aula. Il nostro voto di coscienza reclamava peraltro un'attenzione e una disponibilità a rompere gli schematismi consolidati. Ieri, al contrario, abbiamo sostenuto in Aula la mozione illustrata dal collega di Gruppo Stefano Ceccanti sulla pregiudiziale d'incostituzionalità. il richiamo ivi presente ad Aldo Moro possiede un monito assai attuale e prezioso sull'accortezza che il legislatore, come sosteneva appunto lo statista democristiano a proposito del secondo comma dell'articolo 32 della Costituzione, non si faccia mai interprete di una logica di onnipotenza, immaginando nel campo della cura di violare i confini dell'umano e del lecito morale. In sé valida, questa lezione sollecita, anche in questo nostro passaggio legislativo, l'assunzione di una diversa ma analoga impostazione prudente e responsabile. In fondo, leggendo in filigrana le diverse posizioni, si coglie uno spirito di unità attorno ad aspetti fondamentali della legge: nessuno vuole l'eutanasia, né viceversa l'accanimento terapeutico; si conviene sulla libertà del cittadino a dichiarare anticipatamente le proprie volontà sul trattamento di fine vita. Ci interroghiamo invece, con alterne e vicendevoli recriminazioni, sulla possibilità d'includere l'alimentazione e l'idratazione artificiali tra le disposizioni attivabili con le suddette volontà. Stiamo parlando di interventi meccanici, che a giudizio di tanti colleghi senatori rientrano comunque nelle pratiche di sostegno vitale alle persone impossibilitate a provvedere normalmente. In virtù del principio di autodeterminazione, si dovrebbe perciò accogliere il diritto alla rinuncia secondo le procedure della dichiarazione anticipata di trattamento. E' solo questo il principio da far valere? Solo questo l'orizzonte entro cui inserire il discorso sulla dignità della vita e conseguentemente sulla dignità della morte? Ebbene, se si radicalizza il contenuto dell'autodeterminazione, fino al punto di fare della libertà il centro della vita solo in quanto essa si presenti come vita degna di essere vissuta, allora si apre nell'ordinamento legislativo e nella stessa percezione morale del Paese un problema di coerenza sull'equilibrio di valori incorporati innanzi tutto nella Carta costituzionale. È per questa ragione

che indica la strada di un'eventuale riduzione, o persino dell'interruzione delle attività di sostegno vitale, allorché tra medici e famiglia venga recepita sulla scorta di precise modalità e procedure definite dalle autorità sanitarie - l'intervenuta grave insufficienza delle funzioni cortico-cerebrali della persona malata. di mettere a fuoco quando e come la somministrazione artificiale di sostanze nutritive non cada, magari inavvertitamente, in una zona assai prossima all'accanimento terapeutico. In questo modo si mantiene fluido il ricorso al sapere scientifico in costante evoluzione e aggiornamento, si conserva immutato il ruolo centrale del personale medico-sanitario, si preserva integro lo spazio di valutazione e il contributo dell'ambiente familiare. Dobbiamo fare uno sforzo perché il senso della laicità non venga sciupato o immiserito, nel delicato articolarsi delle sovrane prerogative parlamentari, sulla base di pure convenienze partigiane. Spetta ai cattolici un sovrappiù di attenzione e di rispetto, dal momento che la traduzione sul piano della prassi politica di valori discendenti dalla dottrina e dalla fede impone loro di distinguere rigorosamente tra convinzioni personali e pubbliche responsabilità. Ciò non significa, ad esempio, che il gesto di De Gasperi più volte evocato, in occasione della famosa "Operazione Sturzo", ovvero la sua manifestazione di autonomia nei confronti della Chiesa di Pio XII, costituisca un paradigma in grado di soddisfare le odierne istanze di libertà e laicità, che chiamano in causa le sensibilità dei democratici e in particolare di quelli d'ispirazione cristiana. È chiaro che la vita politica, dalla tattica elettorale alla gestione delle alleanze, rientra a pieno titolo in una sfera di competenza su cui nulla può e nulla deve l'interferenza della Chiesa. Ma il modo in cui si assume l'onere di comporre i valori fondamentali operanti in un contesto religioso con il pluralismo di una società non più descrivibile come *naturaliter* cristiana, è un'operazione più incerta e complicata. A ben vedere la maggiore insidia, sempre attiva nella storia del cattolicesimo politico, è quella di scambiare l'onere della laicità con la pretesa della verità, ovvero con l'esorbitante ambizione di tracciare sul terreno della prassi una versione più raffinata, e quindi più adeguata, della posizione ideale dei credenti. Con il rischio, pertanto, di compiere a rovescio un'invasione di campo: insegnare alla Chiesa ciò che deve dire e come deve dirlo. la nostra discussione ci porta tanto facilmente a debordare da una linea di cautela e di equilibrio, abbiamo bisogno di attenerci ad un codice di profondo realismo. Se il Parlamento troverà la forza di legiferare con il conforto di una larga maggioranza, non coincidente con quella di Governo, dobbiamo essere certi che il Paese ne trarrà solo giovamento. Sarebbe invece azzardato escludere che l'esasperazione di una disputa dai contorni nuovamente ideologici non spinga l'opinione pubblica a maturare un sentimento di delusione sulla capacità della politica di sciogliere i nodi più intricati di questo concitato e decisivo confronto sul potere, nonché sui limiti della legge di fronte alla libertà di ogni cittadino.

onorevoli colleghi, ho chiesto di prendere la parola per intervenire su un tema così spinoso e così delicato perché era stato posto in discussione in quest'Aula il problema il problema se fosse opportuno un intervento normativo del legislatore su temi così complessi come quelli che noi ci apprestiamo a normare. Credo sia assolutamente indispensabile mettere in rilievo come il silenzio del diritto su questo tema sia stato rotto non tanto dal disegno di legge al nostro esame ma, soprattutto, dal progresso della scienza e della tecnica. Non avremmo parlato così a lungo del caso Englaro se i progressi scientifici non avessero consentito interventi e terapie salvavita nei riguardi della vita umana. Sappiamo che le grandi codificazioni civili che hanno tutelato e cercato di tutelare le persone sin dal 1800, sin dal Code Napoléon, avevano messo in rilievo la tutela della persona, sia quale espressione psicofisica che quale soggetto di diritti. Il codice vigente - che risale ai cittadini vivi, a coloro i quali respirano, la capacità giuridica, mentre quello precedente del 1865 stabiliva che questa capacità fosse attribuibile ai soggetti nati e sani. sani. Credo che l'intervento del legislatore in questo ambito, rompendo il silenzio delle leggi naturali, sia dovuto soprattutto al fatto che due grandi eventi che coinvolgono la persona umana e la scienza (la nascita e la morte) sono oggetto di medicalizzazione, di interventi da parte del personale sanitario. Questi due eventi, cioè, non avvengono più secondo il destino, secondo il caso, ma anche attraverso interventi terapeutici. allora sottolineare come l'intervento normativo che ci apprestiamo a porre in essere debba tener conto dei confini normativi che qui sono stati richiamati a livello costituzionale da illustri colleghi, ma che a mio giudizio non hanno posto in rilievo fino in fondo i confini guida entro cui noi ci possiamo muovere. In realtà, se approfondiamo bene i contenuti della nostra Carta costituzionale, ci accorgiamo che i binari fondamentali di questo percorso

Credo che la dignità umana rappresenti, quindi, nel nostro percorso giuridico e normativo - perché di questo si tratta - non solo l'espressione di una visione anche trascendentale, in cui io credo (l'uomo creato ad immagine e somiglianza di Dio), ma soprattutto il riflesso dell'ideologia liberale che pone l'uomo e la persona umana al centro di un sistema di tutele. Se così non fosse, noi non saremmo qui a discutere su quali siano i limiti e le libertà che sono state richiamate dal relatore e dal senatore Saccomanno, sul fatto che appare davvero implicito il rilievo che la vita umana costituisce il presupposto delle libertà fondamentali, non dovevamo certo richiamare il giusnaturalismo dell'articolo 2 della nostra Costituzione, in forza del quale la Repubblica garantisce e riconosce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Ma soprattutto il diritto alla vita costituisce il nucleo essenziale di quella tutela della persona umana di cui i Padri costituenti hanno sottolineato, con capacità espressive, nell'articolo 32, il fondamentale elemento di tutela della dignità. Quando in quest'Aula è stato evocato che i trattamenti sanitari non possono essere somministrati se non in base alla legge, non si sottolineava altro che il principio delle Costituzioni novecentesche,

costituirà un corpo normativo nel nostro ordinamento, in cui sono tracciate le linee essenziali di questo percorso culturale e politico cui sono giunte le culture occidentali europee che si radicano - lo voglio ripetere qui - nella cultura giudaico-cristiana dell'Occidente, si sottolinea che i trattamenti sanitari non possono essere seguiti se non con il consenso dell'interessato, che c'è un divieto al mercato del corpo o degli organi, che c'è un divieto di eugenetica di massa e che c'è un divieto di clonazione riproduttiva, questi sentieri ci portano a sostenere che la dignità umana rappresenta il centro d'imputazione di tutela, non solo delle Costituzioni, ma di tutta la cultura giuridica, politica e sociale dell'Europa occidentale.

dell'alimentazione, si può ammettere che una persona possa morire, credo colpisca questo bene fondamentale che è la protezione della dignità umana, che nel nostro ordinamento è un bene costituzionalizzato. Non è un caso, cari colleghi, che la Grundgesetz, la Costituzione tedesca, inizi con il sottolineare, all'articolo 1, che la dignità umana è inviolabile. Quando in quest'Aula alcuni colleghi hanno sottolineato l'intervento della Corte Suprema degli Stati Uniti o della House of Lords del Regno Unito, non hanno bene inquadrato che il nostro livello di tutela è in una fase molto più avanzata rispetto a quegli ordinamenti. La nostra fase di tutela e il pieno rispetto della Costituzione nel nostro Paese esigono che la vita umana sia tutelata fino in fondo, fino all'ultimo impulso, fino all'ultima speranza di vita, perché questo è quello che costituisce il perno essenziale non solo di una diversità degli ordinamenti giuridici, ma di un diversità del percorso culturale e valoriale della nostra civiltà occidentale. Sono orgoglioso di essere stato eletto in Parlamento, di intervenire in Aula. Ringrazio il collega relatore e tutti coloro i quali si sono prodigati per tutelare la dignità della persona umana con questo provvedimento normativo. Sono convinto che dovremo tornare su questi temi perché, come diceva Günter Andersen nel 1953: "L'uomo ha spostato le sue frontiere sempre più avanti, per cui il rapporto tra il naturale e l'eterointegrazione della scienza, quindi l'ibridità della condizione umana, si è sposata ancora sempre più avanti".

Signora Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, sono due le ragioni per le quali sono profondamente contrario a questa legge: una piccola ed una grande. La ragione piccola è che questa legge, a mio parere, è è scritta ancora male. Vi sono nel testo contraddizioni, incertezze, definizioni normative che potrebbero essere superate da un lavoro di emendamenti e forse dal compimento della discussione che stiamo qui realizzando. Faccio qualche ad esempio: all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, si dice che la legge garantisce la partecipazione del paziente all'identificazione informata e consapevole delle cure mediche più appropriate. E' una espressione francamente inaccettabile. Non tocca al paziente né fare la diagnosi né identificare le cure mediche più appropriate: il paziente non ha ovviamente le competenze professionali proprie del medico, né ha la sua responsabilità professionale. Tocca, invece, al paziente il diritto di essere informato dal medico della pienezza della sua valutazione, della diagnosi e della proposta terapeutica, dei rischi delle alternative e dunque a quel punto esprimere un consenso informato. Possibile che dobbiamo introdurre un principio così mal scritto all'articolo 1 per correggerlo all'articolo 2, dove al comma 2 si dice appunto che l'espressione del consenso è preceduta appunto da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente, in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto dal medico? A cosa serve questa contraddizione ? A far divertire i giudici quando si occuperanno di questa legge? Si potrebbe correggere. Ma non è l'unica cosa che a me sembra che non funzioni. All'articolo 3, colleghi - siamo in discussione generale sulla legge - colpisce il fatto che nella dichiarazione anticipata di trattamento si dice al comma 2 che il soggetto dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica. Il soggetto, il cittadino deve prendere le proprie valutazioni e decisioni in conformità col codice deontologico dei medici? E perché allora non anche di quello degli infermieri? O delle decisioni e del codice deontologico dell'ordine degli avvocati? E quando ci sarà, magari, anche quello degli idraulici? Il cittadino è soggetto alla legge. I medici eleggono i loro rappresentanti negli ordini e definiscono i loro codici deontologici, che valgono per i medici, non per i cittadini. Ma che norma è che norma è quella che stabilisce che il cittadino deve essere subordinato al codice deontologico di una categoria professionale? Davvero continuo a non comprendere cos'è questa legge:

Glielo può dire un amico. Gli chiede: dammi una valutazione di quello che ha pensato questo signore. Serve una legge, un dibattito del Paese, una discussione come questa per arrivare alla grande conclusione che le scelte libere del paziente saranno valutate dal medico? Ma che razza di medico è se neanche le valuta? Davvero non capisco di che razza di testo di legge stiamo parlando, in presenza di contraddizioni che a me sembrano enormi. Non basta; all'articolo 7, comma 5, c'è scritto (ed anche questa mi sembra una una contraddizione) che nel caso di controversia tra il fiduciario e il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio di medici: e dagli a mettere neuropatologi, neurofisiologi, neuro questo e quell'altro. Dopodiché, il parere di questo collegio non è vincolante per il medico. Bene, avranno bisogno di un consiglio per poi decidere come gli pare! Poi, però, leggo, all'articolo 8, che lo stesso parere che non è vincolante per il medico, lo è invece per il giudice tutelare. Ma chi ha scritto questa norma? Un collegio che dà un parere, che non è vincolante per il medico curante, e invece il giudice tutelare deve esprimere un'opinione ad esso conforme? A me sembra anche questa una norma che porta a chiedersi: ma è possibile che il Popolo della Libertà non abbia più un giurista che possa guardare questi testi?

Si è discusso a lungo di tale aspetto. Stamattina abbiamo avuto una lezione dal senatore Nania, che ci spiegava che il diritto alla vita è inviolabile e indisponibile

le coste, le foreste demaniali, le spiagge. Quelli sono beni non disponibili, e francamente la mia vita vorrei che non fosse considerata un bene patrimoniale dello Stato non alienabile. Vorrei che fosse considerata, come dice la nostra Costituzione, un mio diritto inviolabile, come inviolabile, secondo l'articolo 13, è il mio diritto alla libertà personale. Anche su questo punto c'è un po' di strana di strana confusione nel testo, così come ci viene presentato dal lungo lavoro della Commissione e dalle decisioni della maggioranza e del relatore. Non stiamo parlando e del relatore. Non stiamo parlando di eutanasia (ho sentito, ieri in particolare, tanta preoccupazione per il rischio di scivolare verso l'eutanasia attiva e passiva), stiamo parlando di un principio di libertà: il diritto di ogni persona di accettare sul proprio corpo trattamenti sanitari che essa ritiene giusti o ingiusti per sé. Questo diritto è mio, non è del mio medico curante, non è dello Stato. In Unione Sovietica i dissidenti venivano mandati nei manicomi di Stato per essere curati; in altri momenti della storia si usava la violenza sulle persone per cambiargli le opinioni; in un Paese civile, in un Paese libero, sul mio corpo si interviene se io ritengo sia giusto farlo e do il mio consenso. Altrimenti, mettetela come vi pare, mettete le norme che volete in questa pessima legge che approverete (ma che sarà respinta dal buon senso degli italiani), quello che voi state facendo è decidere con questa legge di legittimare la violenza sulle persone: la scelta di usare la forza contro le persone che non vogliono quel trattamento sanitario. Francamente, rispetto all'ultimo intervento che ci decantava la dignità della persona umana, io, che credo fortemente nella dignità della persona umana e che credo che a fondamento di essa ci sia appunto la libertà, non vorrei che fosse usata violenza contro di me. Per le migliori intenzioni di questo mondo, per i migliori stati di coscienza e di scienza del medico curante, non vorrei che contro la mia volontà venisse usata violenza. Questo è il punto di questa legge. Questa è la ragione del dissenso così forte che si è espresso in quest'Aula. Questa è la ragione perché questa legge obbedisce ad una bandiera di principio, alla voglia di affermare un potere dello Stato ed anche, forse, alla voglia di riaffermare una concezione paternalista del medico che decide del destino dei suoi pazienti e non c'è quel coraggio di pensare che l'unica grande prova della dignità e dello straordinario valore di ogni vita umana, sta proprio in questo segreto straordinario che è la libertà*.

credo che il dibattito di questi giorni confermi un aspetto importante, ossia che già da diversi anni, da quando è stata presentata la prima proposta di legge sulle questioni di fine vita, il livello del confronto è sempre stato difficile. Lo sarà ancora oggi, se volessimo dare delle risposte univoche, da una parte al principio dell'indisponibilità della vita, che deve comunque essere strettamente legato agli altri valori e principi inviolabili (la libertà, la dignità,

che deve saper rispettare l'esigenza di tutela del proprio corpo e della propria esistenza anche rispetto a invadenze non accolte dalla nuova tecnologia medica. Quali che siano i sentimenti, le convinzioni ideologiche e il credo religioso di ciascuno di noi, tali considerazioni e le valutazioni che ne dovranno seguire, in questo dibattito e nell'approvazione o meno della legge, non potranno limitarsi al solo ambito dei princìpi morali, ma dovranno entrare nel vivo di questioni giuridiche ben precise e avere la sola ambizione di dare un fondamento giuridico a condizioni particolari della nostra vita - perché di questo si sta parlando e non di Alzheimer o di disabili senza che i sostenitori dell'una o dell'altra tesi debbano avere la pretesa di essere gli unici interpreti della Costituzione. Il compito dei legislatori, il nostro compito, non è di fare soltanto una legge nell'intento attualizzato e comprensibile di colmare presunti e, a volte, anche pericolosi vuoti legislativi, bensì di realizzare una buona legge che, per essere giusta, deve essere in grado di riaffermare nel nostro ordinamento giuridico, nel rispetto del pluralismo, la centralità della persona umana nella molteplicità delle sue esigenze e delle sue manifestazioni esistenziali. Su questa premessa, riteniamo che il punto importante da cui partire sia il seguente: la dichiarazione anticipata di trattamento, oggetto del provvedimento legislativo altro non è che lo strumento con cui estendere il consenso informato (un diritto ormai acquisito, a meno che non vogliamo mettere in discussione anche questo)

tale diritto, ossia che la volontà individuale, adeguatamente informata, sempre suscettibile di ripensamento, costantemente assistita dal rapporto terapeutico e da una rete di relazioni familiari e sociali, può e deve assumere la decisione che riguarda le cure da ricevere, sempre e anche nel caso si perdesse la facoltà di decidere. Nessuna autorità può e deve sostituirsi a tali decisioni e decidere senza tenere conto della volontà del malato. Ad affermare ciò sono la Carta costituzionale, la Convenzione di Oviedo, l'intera giurisprudenza italiana. Questo, a mio giudizio, è il punto da cui partire, su cui penso possa esserci una serena convergenza. evidente che, nonostante i tentativi di mediazione, il dibattito intorno alla presente legge è più o meno fermo su due punti: i limiti dell'accanimento terapeutico (articolo 1, lettera *f)* del testo proposto dalla Commissione) e se esso include o meno l'idratazione e l'alimentazione forzata (articolo 3, comma 6).Vorrei fare alcune considerazioni sul primo dei due aspetti. «Per il medico e i suoi collaboratori non si tratta di decidere della vita o della morte di un individuo. Si tratta semplicemente di essere medico, ossia di interrogarsi e decidere in scienza e coscienza la cura rispettosa del vivere e del morire dell'ammalato a lui affidato. Questa responsabilità non esige il ricorso sempre e comunque ad ogni mezzo. Può anche richiedere di rinunciare a dei mezzi, per una serena e cristiana accettazione della morte, che è inerente alla vita. Può anche voler dire il rispetto della volontà dell'ammalato che rifiutasse l'impiego di taluni mezzi». Sono parole, concetti, contenuti importanti, che si lasciano apprezzare per la loro straordinaria laicità e che poi scopriamo essere presenti nella Carta degli operatori sanitari, pubblicata nel 1996 dal Pontificio Consiglio per la Pastorale della salute. La Carta, che afferma quanto riportato, è tuttora compresa tra i documenti della Pontificia Accademia per la vita e si colloca, quindi, all'interno del pensiero cristiano. Non spetta a noi l'ambizione di fare pronunciamenti morali o, peggio, di voler alimentare un conflitto politico-parlamentare sul piano dei principi. Se vogliamo restare fermi alla nostra funzione legislativa - perché è questa alla quale siamo chiamati - vi è un'altra questione a cui dovremmo dare una risposta: in caso di controversia sulle decisioni di cure mediche tra medico e paziente, perché mai dovrebbe prevalere, alla fine, la decisione del medico? A questo quesito risponde, non dico con buon senso, ma secondo scienza e coscienza, l'articolo 38 del codice deontologico dei medici dove si legge che «Il medico deve attenersi, nell'ambito della autonomia e indipendenza che caratterizza la professione, alla volontà liberamente espressa della persona di curarsi e deve agire» - - «nel rispetto della dignità, della libertà e autonomia della stessa». Vengo ora alla seconda questione, perché i progressi della scienza, inimmaginabili sino a pochi anni fa e inimmaginabili ancor di più tra qualche anno, ci chiedono che nell'orizzonte della difesa della dignità umana deve essere affrontato anche il tema della nutrizione e idratazione artificiale. Non voglio ricordare espressioni forti, che offendono la nostra coscienza, come quella che nel nostro Paese non si può morire di fame e di sete, che non aiuterebbero la ricerca di una legge giusta per tutti, ponendo, al contrario, vere e proprie barriere che di fatto svuoterebbero dal di dentro e in partenza lo spirito del testamento biologico, lo spirito di questa legge. Voglio anche comprendere le ragioni di parte, ma non condividere la posizione autorevole espressa alla stampa da un sottosegretario di Stato, l'onorevole Roccella, quando sostiene, in una interpretazione del tutto personale dell'articolo 32 della Costituzione, che «in Italia la libertà di cura, nella interpretazione dei magistrati, è scivolata verso il diritto a morire». Mi limito semplicemente a confutare alcune argomentazioni, pure autorevoli, come quelle espresse dal parere del Comitato nazionale di bioetica nel 2005 che ritenne, con un voto a maggioranza e non unanime, che la richiesta di sospensione del trattamento di alimentazione forzata si configurasse in una vera e propria eutanasia omissiva. Sono sensibilità e posizioni rispettabilissime che però, per noi, non possono andare in contrasto con le acquisizioni di gran parte della comunità medico-scientifica internazionale, che considera la nutrizione artificiale un trattamento medico e, quindi, come tale, non può essere attuata in presenza di una volontà contraria del paziente. Lo ha ribadito, tra gli altri, in modo chiaro, il presidente della Società italiana di nutrizione artificiale professor Muscaritoli, quando ha dichiarato che nutrizione e idratazione artificiali vanno considerate trattamenti medici e, come tali, da non somministrare indiscriminatamente e indipendentemente dallo stato di coscienza. Noi rispettiamo sensibilità e posizioni diverse, ma queste non possono andare in contrasto con i fondamenti deontologici della professione medica, dove all'articolo 53 del codice deontologico si afferma che «quando una persona rifiuta volontariamente di nutrirsi se è consapevole delle possibili conseguenze della propria decisione, il medico non deve assumere iniziative costrittive né collaborare a manovre coattive di nutrizione artificiale nei confronti della medesima, Noi rispettiamo sensibilità e posizioni diverse, come pure la sensibilità che emerge in gran parte del mondo cattolico, che ha saputo esprimere rispetto per le coscienze individuali, nell'accogliere

si accetta di non poterla impedire". È un concetto completamente diverso, che non ha nessun riferimento a derive eutanasiche. Se poi

Noi abbiamo questa grande responsabilità perché su questa legge, se dovesse mancare l'intesa convinta e comune su temi tanto delicati, non si rischia che il Paese si spacchi in due ‑ come è stato detto ma che l'unica spaccatura sia tra il sentire comune del Paese e chi è chiamato a rappresentarlo*. Signora Presidente, onorevoli senatori, signor Sottosegretario, nel nostro Paese è in atto un dibattito che investe le coscienze, che tocca le nostre sensibilità e che coinvolge nel profondo delicati problemi etici. Oggi siamo dinanzi alla possibilità di compiere un piccolo passo avanti per colmare quel vuoto legislativo, che ha posto all'attenzione dell'opinione pubblica (forse negli ultimi tempi in maniera anche troppo coinvolgente) il problema del fine vita. Lo smarrimento non è stato solo quello percepito in generale ma tutti noi ci siamo trovati impreparati, quasi incapaci di dare risposte giuste a interrogativi che vanno oltre la dimensione politica *tout court*. Il dibattito ha coinvolto tutta la società italiana e in primo luogo il Parlamento, che è stato accusato di non aver mai affrontato fino in fondo il problema. In passato, la tentazione di rimandare e di continuare a discutere ha prevalso e ha lasciato il nostro Paese senza una normativa, recepita invece - e da tempo - in altri Paesi europei. Recuperare il tempo perduto rappresenta un'esigenza imprescindibile. Il caso di Eluana Englaro ha determinato un'onda emotiva forte che tanti, su versanti opposti, hanno tentato di cavalcare. Io credo sia invece utile che il legislatore sappia mantenere un giusto distacco, il che non significa affrontare la tematica con freddezza o indifferenza. C'è la necessità di una legge costruita con l'apporto di tutti e che non chiuda le porte a proposte o modifiche di buon senso. Mettiamo da parte le incomprensioni e le divisioni che ci hanno accompagnato sino ad oggi. È, questo dibattito nell'Aula del Senato, la prima occasione per riavvolgere e mettere in soffitta quel filo spinato che ci ha diviso fra partiti e nei partiti. Tutti sentiamo la necessità di una legge largamente condivisa e, forse, attraverso il confronto serio ed approfondito, sarà possibile pervenire ad un risultato soddisfacente. Una legge, anzi la legge, se vuole difendere il bene della vita, lo deve fare tutelando la vita in tutte le sue fasi. Difendere una vita è curare chi chiede di essere curato, ma anche cercare di convincere chi non vuole essere curato a desistere dall'idea di soccombere al male. Allo stesso modo e per le stesse ragioni, difendere la vita non è obbligare alla cura chi decida consapevolmente di sottrarsi. Difendere la vita, perciò, non significa "costringere alla vita". In casi come questi, etica e politica devono trovare un terreno di incontro che diventi una base di partenza per coniugare la conoscenza scientifica, il sapere giuridico e l'azione legislativa. Onorevoli senatori, ricordo a tutti noi che la vita non è qualcosa. È sempre qualcuno, è un individuo! È da questa considerazione, prima ancora che dalle norme, che discende il principio di cura e terapeuticità, che enuncia il dovere morale del rispetto del corpo e della tutela della salute e della vita propria ed altrui. Ognuno di noi ha delle idee su questo tema. quindi, di dividerci in laici e cattolici, in buoni e cattivi, in chi difende la vita e chi no, ma si tratta di fare uno sforzo e di evitare radicalizzazioni che non portano da nessuna parte. Non dobbiamo, insomma, alimentare una sorta di bipolarismo etico, ma dobbiamo essere pronti a trovare, anche con fatica, una sintesi politica che non perda di vista la sfida che abbiamo davanti, che è quella del pluralismo, della capacità di rispettare ogni idea tenendola nella giusta considerazione anche tramite una mediazione che, ovviamente, non prescinda dal rispetto della vita e della dignità della persona umana. Non possiamo negare che questi sono valori condivisi, appartenenti non solo ai cattolici ma espressione anche di un patrimonio laico. Mi piace ricordare al riguardo il monito di Zaccagnini che sottolineava: "Siamo in politica non in nome della fede, ma a causa della fede". È chiaro che una qualsiasi legge - figuriamoci su una materia tanto delicata - non può codificare gli ambiti etici e tutti gli aspetti valoriali di un sistema, ma certamente può essere un punto di partenza su cui trovare una convergenza o almeno uno spunto di riflessione più ampio e costruttivo. Non credo sia il momento, infatti, di accentuare fratture e divisioni, di proporre un clima di spaccatura netta tra diverse visioni. È indispensabile, invece, lasciare al Parlamento le chiavi della discussione e della riflessione. Il testo in esame è sviluppato da un intenso confronto politico

Per questo, credo che la strada maestra sia quella del dialogo tra tutti coloro che hanno a cuore l'obiettivo di rendere questo testo migliore di come è entrato in quest'Aula. Prima di tutto non dobbiamo perdere di vista i princìpi costituzionali su cui non si può derogare. La nostra Costituzione dimostra con estrema chiarezza che l'ispirazione cristiana può e deve divenire patrimonio laico della Repubblica. L'articolo 32 afferma che "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti". comma esplicita chiaramente il principio di base che deve ispirare l'intera legge: "Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana". C'è, insomma, già nella Costituzione la libertà di scegliere a quali trattamenti sanitari sottoporsi e a quali non sottoporsi. Non possiamo dimenticare che altri punti fermi sono stati acquisiti dal Paese. Il consenso informato è una grande conquista etica che copre l'intera vita del soggetto garantendo, comunque, il diritto di uscita dalle terapie ed il rifiuto delle cure. Si tratta di appropriarsi della decisione su "se e a quali cure sottoporsi". Il vincolo dell'autodeterminazione è la corretta informazione che diviene tanto più efficace quanto più si terrà conto delle specificità che ogni situazione concreta presenta. Perché quell'alleanza terapeutica, che tutta la legge non deve mai perdere di vista, richiede la partecipazione attiva del paziente sulle scelte che lo riguardano, attraverso uno scambio continuo ed approfondito di informazioni con il medico. Per tale motivo, l'inserimento del consenso informato e l'autodeterminazione tra gli aspetti cardine del disegno di legge rappresenta veramente una nostra piccola vittoria: sono princìpi che trovano, nel testo in esame, concreta dignità. Per entrare più nel dettaglio, non posso non esprimere, invece, dubbi e perplessità in riferimento alla lettera *b)* dell'articolo 1 del testo che "riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e della scienza". A me sembra un'affermazione generica, innanzi tutto perché non si capisce quale sia l'interesse della società e della scienza, chi lo decida e chi lo misuri; in secondo luogo, perché non è chiaro cosa s'intenda con la dicitura "in via prioritaria". Non dobbiamo mai dimenticare, infatti, che la dignità dell'uomo è un diritto assoluto e non solo prioritario rispetto agli altri. Su due punti, che hanno in questi giorni acceso il dibattito politico, voglio essere il più possibile chiara. Al riguardo, desidero che non si confonda la mia personale visione dalla posizione del partito. Un partito moderno come il Partito Democratico deve potere accogliere nel suo interno diverse opinioni, in particolare su temi delicati come quello del fine vita. E questo, colleghi senatori, non è segno di debolezza, ma è una ricchezza. Il primo punto è quello dell'idratazione e della nutrizione. Li considero un sostegno vitale e quindi non atto di accanimento terapeutico, elemento per cui verrebbe meno il dovere di cura. Infatti, l'idratazione e la nutrizione artificiali non possono essere considerati atti terapeutici, volti cioè al miglioramento dello stato di salute del soggetto, ma semplicemente atti il cui unico scopo ed effetto è quello di mantenere in vita un paziente, assicurandogli la soddisfazione dei propri bisogni primari. Recentemente, la stessa Cassazione, definendo la nutrizione e idratazione artificiali come trattamento sanitario, ha dichiarato che "questo non costituisce oggettivamente una forma di accanimento terapeutico, ma rappresenta piuttosto un presidio proporzionato rivolto al mantenimento del soffio vitale". Detto ciò, sono ugualmente convinta esistono però casi eccezionali dove ipotizzare la sospensione dell'idratazione e della nutrizione è corretto. Ed è proprio su questo punto, colleghi senatori, che chiediamo alla maggioranza di non chiudere la porta al dialogo, ma di lavorare insieme. Il secondo punto di approfondimento è quello relativo al comma 7 dell'articolo 3, nel quale si dice che "la dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario". Insomma, nel testo, il rilievo delle dichiarazioni viene riconosciuto solo se il soggetto è in uno stato vegetativo. formula non può vederci d'accordo, perché rischiamo di licenziare una legge *ad personas*, cioè rivolta solo a quelle poche (2.000-2.500) persone che si trovano attualmente in questa condizione. persone che non sono neppure in grado di sottoscrivere una dichiarazione di intenti, per cui siamo di fronte ad una norma che in concreto oggi non tutela nessuno. Vorrei concludere osservando che una legge di questa portata non può non contemplare il capitolo delle terapie contro il dolore. Tramite le cure palliative, ci ci si propone proprio di accompagnare il paziente nel tragitto verso la guarigione o, nella peggiore delle ipotesi, verso la morte. Partendo dal presupposto che non soffrire deve essere un diritto, mi auguro che non si dimentichi l'impegno che è stato preso anche in Commissione, affinché venga introdotta nel nostro ordinamento una seria disciplina sulle cure palliative. In definitiva, colleghi senatori, abbiamo oggi ancora una volta una grande responsabilità nei confronti dei nostri concittadini. Dobbiamo cercare di evitare di mettere in scena una versione aggiornata della disfida tra guelfi e ghibellini. Il nostro compito è quello di scrivere una buona legge, che aiuti persone che soffrono, i loro familiari e i medici che li hanno in cura ad affrontare i terribili momenti della fine della vita. È a questo dovere che dovremmo ispirarci sempre. Per parte nostra, confermo a tutta l'Assemblea la sincera volontà di dialogare e confrontarci, per approvare un testo il più possibile condiviso. Grazie, signora Presidente, grazie, onorevoli colleghi senatori.

Onorevole Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, consegnerò il testo scritto del mio intervento, però utilizzerò ugualmente il tempo che mi è concesso, proprio

lavori della Commissione, che non posso dire distratta - e che quindi non viene dalle valutazioni che, anche ieri, ho potuto esprimere in risposta alla richiesta di pregiudiziali

«C'è una categoria di diritti indisponibili che noi giuristi conosciamo - forse la apprendiamo il primo anno di giurisprudenza - ed il primo di tali diritti è il diritto alla vita. Conseguenze Conseguenze di questa indisponibilità e di questa impostazione abbastanza scontata sono il divieto e l'illiceità dell'eutanasia, e non solo dell'eutanasia, ma anche di ogni intervento sanitario che comporti la soppressione della vita, nonché l'incostituzionalità di una legge ordinaria che invece li ammettesse anche indirettamente». Non era, quindi, un pensiero peregrino né quello di chi ha formulato il testo di sintesi delle altre proposte presentate, né quello di chi in questi giorni, sia pure nel centrodestra, si è affacciato ad ipotesi di difesa della vita e della dignità della stessa correlate ad un momento costituzionale importante e ad una riflessione indubbiamente alta.

elementi di riflessione importanti, di fronte ai quali credo che ci siamo interrogati positivamente, impegnandoci tutti. È mancata forse da parte della maggioranza la sensibilità per affrontarli in modo giusto? Non abbiamo forse compreso la forza della prima parte di quell'emendamento? In essa, non solo nella mozione espressa in quest'Aula dal Partito Democratico, ma in Commissione, con l'autorevolezza della presidente Finocchiaro, veniva a consolidarsi la scelta che idratazione ed alimentazione, senatore Cosentino, sono sostegno vitale e si cercava un labile appiglio, non so quanto solido, riuscire a trovare delle eccezioni. Noi abbiamo difficoltà ad accettare eccezioni. Abbiamo difficoltà a pensare che la vita abbia un suo valore in base agli aggettivi che ci sono intorno. Per noi la vita è vita, va salvaguardata, resa preziosa e, nel momento in cui è ferita, aiutata. Certo i momenti di solitudine sono probabilmente quelli che poi fanno prendere le scelte sbagliate.

dovrà fermarsi, riprendersi in carico quella persona e cominciare a vivere in simbiosi ed in sinergia per una vita che si vuole difendere e che non si vuole lasciare. Certo, le cure palliative affinché siano aiutati. Le cure per loro e le famiglie. C'è un ordine del giorno che abbiamo proposto tutti. Molti sono i partiti che lo hanno firmato. il PD, che probabilmente ne presenterà un altro. Certamente c'è un impegno a lavorare in questo senso, un impegno condiviso, con un documento firmato in Commissione anche dal PD che accettava che la Camera si interessasse non voglio dilungarmi oltre sul punto. I tre concetti principali di questa legge sono tre grandi concetti, senatore Cosentino. Il consenso informato è la prima volta che viene normato. C'è una norma chiara che impone al medico di informare. Possiamo poi giocare, ridicolizzare la norma, che si può migliorare per come si scrive, ma sappiamo che da oggi non sarà un foglietto da firmare occasionalmente e di sfuggita prima di entrare in sala operatoria. C'è una norma chiara, precisa e positiva

per una giusta lettura. Sembra poco? Abbiamo detto, e lo scriviamo, non dal Comitato di bioetica, non da altro, pur confrontandoci con la coscienza e con il codice di deontologia medica, che l'accanimento terapeutico o il cosiddetto accanimento clinico è certamente qualcosa che non esiste nella possibilità delle cure previste nello Stato italiano. La Repubblica dice che quelle possono e devono essere bandite. non è una conquista importante trovare una norma positiva in proposito? Non stiamo parlando di leggi per i credenti. In quel che dico ci sono leggi laiche e organizzative per uno Stato che deve produrre un determinato effetto. Questo anche quando parliamo di idratazione e alimentazione. Abbiamo scelto tutti

Vorrei che le norme potessero stabilire che quando uno è morto non va assistito oltre. Questa è la norma su cui riteniamo di difendere la nostra legge, ma non con un muro, perché può essere migliorata. L'abbiamo sempre detto, ribadito e praticato. Può essere migliorata con il concorso di tutti, certamente per il bene di una grandissima comunità e non solo di poche persone. *(Applausi